come gli onorevoli senatori sanno, nella notte tra il 3 e il 4 novembre diversi parlamentari dell'HDP, la terza formazione parlamentare turca, tra cui i due copresidenti Demirtas e Yuksedag, sono stati arrestati e tuttora dieci tra questi parlamentari sono trattenuti in carcere. Domani gli avvocati dei due copresidenti presenteranno ricorso alla Corte costituzionale turca contro il loro arresto; nel frattempo la sede di Ankara dell'HDP è ancora chiusa. Subito dopo questi arresti ho espresso a nome del Governo la nostra viva preoccupazione per un fatto che deriva peraltro dalla decisione nel maggio scorso, approvata a maggioranza, di abolire l'immunità parlamentare nel Parlamento turco. Ho espresso la preoccupazione del Governo e la stessa è stata ribadita nei giorni successivi dal nostro ambasciatore ad Ankara. Certamente conosciamo il contesto in cui oggi si trova la Turchia; conosciamo la gravità del tentativo di colpo di Stato che c'è stato lo scorso 15 luglio. Io stesso ho visitato Ankara e sono stato, tra l'altro, nella sede del Parlamento in cui sono evidenti i segni del bombardamento che è avvenuto quella notte, così come sono evidenti i segni di proiettili e di missili sia nella residenza di Erdogan sia negli uffici di alcuni Ministeri. Conosciamo anche la frequenza degli attacchi terroristici sia del PKK che di Daesh, di cui la Turchia è oggetto, e non abbiamo mai mancato di esprimere la nostra solidarietà di fronte a questo tentato *golpe* e di fronte agli attacchi terroristici ad un Paese che - tutti sappiamo - oltre a essere membro della NATO, è un Paese chiave nella Regione per l'andamento di diverse crisi: dalla Siria alla Libia, all'Iraq. Deve essere, però, molto chiaro che questo contesto, la cui serietà non ci sfugge, non può giustificare in alcun modo gli arresti dei *leader* di una grande forza di opposizione parlamentare. Arresti che seguono, peraltro, quelli effettuati nelle ultime settimane, anche di giornalisti, con la chiusura di testate giornalistiche;

è proprio la possibilità o meno che si attivi un dialogo, un percorso politico, teso a tentare di risolvere la questione curda non attraverso un confronto militare ma attraverso la ricerca di una soluzione politica. Ebbene, l'interlocutore ovvio di questo tentativo è proprio l'HDP, ovvero il partito che è stato oggetto di queste operazioni. Anche dall'incontro che ho avuto ad Ankara con il *leader* del partito Demirtas alla fine dello scorso anno avevo tratto esattamente questa convinzione, e cioè che lì ci fosse un sentiero. Qualcuno ha parlato in questi anni di paralleli un po' audaci con la situazione irlandese, ma comunque senza dubbio c'era lì una distinzione tra una scelta terroristica e militare e la scelta di una forza di opposizione parlamentare. Rivolgere nei confronti di questa forza parlamentare un'operazione come quella degli arresti ovviamente chiude questa prospettiva ed è molto grave: io credo che questo sia avvenuto. Non è un caso che a condannare l'operazione siano stati anche gli altri partiti di opposizione parlamentare, e non solo, come ovvio, l'HDP oggetto di questi arresti. L'altro ieri ne abbiamo discusso con i colleghi Ministri degli esteri europei al Consiglio affari esteri a Bruxelles, ribadendo due valutazioni: la prima, che questi arresti sono inaccettabili; la seconda, invitando le autorità turche a ritornare al più presto possibile ad un un funzionamento, per quanto limitato e parziale, delle regole di base dello Stato di diritto. Molto si discute - lo abbiamo fatto anche a Bruxelles - delle evoluzioni in generale dei rapporti tra Turchia e Unione europea. Sapete, onorevoli senatori, che il nostro Paese è stato negli ultimi quindici anni - perché è una storia che non è nata ieri - costante sostenitore di un percorso tra Unione europea e Turchia, nella convinzione che questo percorso fosse, in quanto tale, utile

il mantenimento di uno Stato laico, sia pure in un Paese a maggioranza islamica; il ripristino di un'autorità da parte del Governo nei confronti delle Forze armate, altra grande questione, per via della tradizione kemalista, aperta nello scenario politico turco; e, per l'appunto, una via negoziale per affrontare la questione curda. Noi abbiamo sempre pensato che il binario di dialogo tra Unione europea e Turchia potesse favorire tutti questi processi positivi. Oggi questo percorso appare sempre più in salita. E appare sempre più in salita - devo essere molto chiaro - innanzitutto per responsabilità delle stesse autorità di Ankara; ma nel momento in cui diciamo questo non dimentichiamo anche le responsabilità europee, perché non sarebbe onesto. Era un negoziato, come si dice in gergo diplomatico, *open* *ended*, ossia non doveva avere necessariamente un traguardo prestabilito di adesione della Turchia all'Unione europea; poteva anche procedere senza dare per scontato che la sua conclusione sarebbe stata, un giorno, l'ingresso della Turchia nell'Unione europea (questo vuole dire negoziato *open ended*). Noi lo abbiamo sempre sostenuto in questo senso. Questa è stata la linea di Romano Prodi e di Silvio Berlusconi negli ultimi quindici anni; purtroppo non è stata la linea di alcuni altri Paesi europei, che hanno semplicemente opposta un «no, mai» alla Turchia. Credo che questo abbia, almeno in parte, contribuito, purtroppo, alle responsabilità che - ripeto - sono prevalentemente, ovviamente, delle autorità di Ankara in merito alla situazione complicata che c'è adesso. Adesso abbiamo in piedi con la Turchia un accordo sulle migrazioni; è discusso ma funziona, nel senso che ha ridotto in modo drastico e senza violazioni sostanziali dei diritti umani

sapete che l'Unione europea adotta 72 criteri, molto precisi e chiari, che difficilissimamente possono essere rispettati oggi dalla Turchia:

delle violazioni che noi abbiamo denunciato. È inutile negarlo, quindi: questo percorso, cominciato tanto tempo fa, per responsabilità delle autorità di Ankara ma anche con il contributo di alcuni Paesi europei, è ormai sempre più stretto e se gli accenni, che ogni tanto si avvertono, di ripristino della pena capitale dovessero tradursi in pratica sarebbe un percorso automaticamente concluso. Infatti, in virtù dei trattati, l'Unione europea non può avere alcuna forma di

al di là di questo, sono gli arresti, sono le decisioni prese in questi mesi e in queste settimane che rendono lo sviluppo di questo itinerario - ripeto - molto impervio e problematico. Ma io dico - e questa è l'opinione assolutamente prevalente nell'ambito dell'Unione europea - che non saremo comunque noi a chiudere formalmente la porta, per una ragione molto semplice. Le regole europee sono molto chiare,

a queste regole e a questi valori noi ci atteniamo. Il fatto che si tratti di un alleato importante e magari di un alleato chiave sul tema delle migrazioni non ci induce assolutamente a rinunciare a queste regole e a questi valori. Sta alla Turchia decidere se andare nella direzione dell'Europa oppure - come sembra in questi mesi e in queste settimane - se proseguire in una direzione opposta. Non saremo noi a sbattere la porta, per una ragione molto semplice: non vogliamo fornire alibi, da questo punto di vista. Se qualcuno vuole assumersi la responsabilità di non proseguire nella ricerca di un rapporto con l'Unione europea, se ne assuma la responsabilità. Noi stiamo alle nostre regole, stiamo ai nostri valori, ma non creiamo alibi per nessuno. *(Applausi Il ritardo nell'inizio della seduta per la mancanza del numero legale mi costringe ad un rispetto rigoroso dei cinque minuti concessi ad ogni senatore, dato che il Ministro deve allontanarsi per altri impegni già programmati. Dichiaro aperta la nuova finestra") *(CoR)*. Onorevole Ministro, mi pare che le sue considerazioni si siano concentrate soprattutto sull'accordo sull'immigrazione, sui criteri europei per la concessione dei visti più genericamente, sul rapporto fra la Turchia e l'Unione europea. Già, ma in base alla sensazione di questi ultimi anni, da questo punto di vista, non mi riconosco molto nella considerazione storiografica di una linea comune Grazie

al matrimonio della figlia di Erdogan (non ancora Presidente del Consiglio) e Romano Prodi (non al Governo ovviamente, ma

Per quanto concerne l'accordo sui migranti, certo per ora sta funzionando. Però il presidente Erdogan ha precisato e sottolineato che, se entro quest'anno non verrà abolito il visto di ingresso per i turchi nell'area Schengen, questo accordo sarà rimesso in discussione. Siccome alla fine dell'anno non manca molto e siccome evidentemente non esiste più, da molti anni, un rischio immigrazione dalla Turchia, è evidente che le procedure Schengen, abolite per gli altri Paesi europei e fatte tranquillamente violare (neanche appannare) per i cosiddetti migranti economici, non possono valere e colpire soltanto turisti ed imprenditori provenienti dalla Turchia. Certo l'Italia - come lei ricordava con orgoglio - ha fatto non bene, ma benissimo ad esprimere a maggio la propria preoccupazione per l'abolizione in Turchia dell'immunità parlamentare. Anzi, da questo punto di vista sarebbe auspicabile un maggior senso critico sulla nostra storia nazionale. Ci avviamo la prossima settimana a ricordare Giovanni Amendola, abbiamo ricordato e ricordiamo spesso Giacomo Matteotti. Dobbiamo ricordare, con analogo disgusto, quando, fra il 1992 e il 1994, alcuni magistrati, poco rispettosi della Carta costituzionale e poco rispettosi della toga che avevano indosso, imposero al nostro Parlamento una giacobina cancellazione di quell'istituto Turchia considerare gli ultimi arresti, quelli cui lei faceva riferimento, una conseguenza indotta dal tentato dal tentato colpo di Stato del 15 luglio. E da allora da questo punto di vista non c'è dubbio che il regime, di fatto presidenzialistico ma di diritto parlamentare (e bisogna ricordarlo), del presidente Erdogan sia oggi un po' un uomo solo al comando della corsa, spesso evocato da cronisti meno intelligenti del collega Zavoli quando seguiva il Giro d'Italia. Se mi è consentita una ultima preoccupazione, che giro al Governo italiano e a quelli dell'Unione europea, è incredibile come si sia sottovalutato che la Turchia viva da un secolo nella sindrome di Sèvres, nel terrore di essere smembrata come territorio. E tutti dimenticano che ci fu dopo Sèvres il trattato di Losanna nel 1923, che costrinse le potenze occidentali a tornare al tavolo negoziale per dare certezza di confini alla Turchia. pur nei diritti, molte volte legittimi, dei curdi è stato "brillantemente" ignorato dalla diplomazia occidentale. Mi riferisco soprattutto al segretario di Stato Clinton e al presidente Obama negli ultimi tempi. Di qui molti errori a catena. *(Applausi dal Gruppo ho ascoltato la sua relazione che, ovviamente, si è svolta in termini molto diplomatici e anche abbastanza generali. A ridosso del cosiddetto *golpe* in Turchia, un autorevole membro di questa Assemblea ebbe modo di rivolgersi io penso che essere troppo avvezzi porti all'assuefazione.

preoccupanti da un bel po' di tempo. Il progressivo abbandono della laicità, indicata storicamente da Ataturk, è in atto da un po'. Già qualche anno fa vi furono degli interventi sull'esercito, anche con dei processi, proprio perché, come lei mi insegna, l'esercito in Turchia è sempre stato il testimone di quella laicità che poteva portare forse a ragionamenti diversi. Come lei sa, storicamente noi non siamo mai stati favorevoli all'ingresso della Turchia in Europa per molti motivi: oltre che valoriali, anche perché riteniamo riteniamo che il ruolo della Turchia debba essere (o poteva essere) svolto in modo diverso in quello scenario. Pochi anni fa, signor Ministro, la Turchia si era posta in una posizione di dialogo duro

non dimenticando di essere anche un crocevia energetico. E questo lo sappiamo benissimo. La preoccupazione, dunque, signor Ministro, non è rivolta unicamente alla Turchia, ma anche al nostro ruolo in quello scenario purtroppo difficile e drammatico. Cosa farà la Turchia con i curdi?

che spero vorrà tenere in considerazione, con la buona volontà di fornire strumenti utili al Governo per potersi orientare a fornire un giudizio in questa circostanza. Il primo fattore che prendo in considerazione è il giudizio, che sembra consolidato, per cui la parabola involutiva della democrazia turca sarebbe un fatto recente. Vorrei ricordare, invece, che il 5 febbraio del 2006 veniva ucciso don Andrea Santoro e, nonostante le testimonianze raccolte dalla magistratura all'epoca dicessero con chiarezza che a ucciderlo fosse stato un uomo adulto adulto penetrato all'interno della chiesa al grido di «Allahu Akbar», venne accusato e si autoaccusò dell'omicidio un ragazzo di sedici anni, Oğuzhan Akdim. Pochi mesi dopo, il 19 gennaio del 2007, veniva freddato con tre colpi d'arma da fuoco alla gola, davanti al giornale «Agos», che aveva fondato e dirigeva, Hrant Dink, un giornalista di origine armena già condannato in Turchia perché aveva scritto, per l'appunto, un libro sul genocidio armeno. Da chi veniva ucciso Hrant Dink? Secondo le testimonianze raccolte, da uomini adulti, ma anche in quella circostanza si accusava dell'omicidio e veniva poi condannato un ragazzo di sedici anni, Ogün Samast, di Trebisonda, la cui presenza all'interno della stazione di polizia di Trebisonda venne resa nota al mondo perché gli ufficiali di polizia fecero ripetute foto con lui prima di consegnarlo alla magistratura. Il 27 ottobre del 2010 la magistratura turca, nell'istituzione della decima Corte amministrativa, condannò il Ministero dell'interno - e quindi gli uomini del KP che lo dirigevano per non avere vigilato su Hrant Dink, che era appunto sotto stretta sorveglianza perché imputato in alcuni processi contro il Governo. Ministro, cosa dicono questi fattori? L'involuzione di un grande partito come il KP è un fenomeno non di oggi, ma è cominciato da molto tempo. Come da molto tempo è cominciata in Turchia la lotta sotterranea tra quel partito e le altre istituzioni dello Stato, che ha come oggetto la contesa per il potere, sul quale il Governo Erdogan da anni ha inserito anche una ulteriore temibile variante: la ripresa di una politica neo-ottomana che ha puntato, ad esempio, a destabilizzare l'Egitto attraverso

e che mira in modo saldo a governare anche l'orientamento di ciò che succede in Libia. Per queste ragioni mi permetto di suggerire al Governo di sollecitare, nell'interlocuzione con la Turchia, la volontà di arrivare nel tempo a una ripresa di consapevolezza della società turca e di sottolineare quanto sia indispensabile un livello adeguato di pluralismo e di governo delle istituzioni per poter essere realmente alla pari nelle istituzioni sovranazionali nelle quali condividiamo responsabilità. Ricordo, per inciso, che le forze armate turche ammontano a 1.181.000 effettivi e che la somma degli effettivi di Germania, Francia e Italia non arriva a questo numero. Mi permetto di concludere ricordando un fatto ulteriore: tutti i giudici che hanno partecipato a quei processi e a quelle sentenze sono oggi in arresto. allieve, gli allievi e i docenti del Liceo classico «Annibal Caro» di Fermo, che stanno seguendo i nostri lavori.

l'odierno dibattito é molto importante, e non solo perché discutiamo di un Paese che ricopre un ruolo fondamentale per gli equilibri tra Europa e Medio Oriente, ma anche perché ci troviamo a discutere di temi importanti, quali la tutela dei diritti umani, l'economia e il confine sempre sottile tra *Realpolitik* e ideali. Parto da questa seconda parte per evidenziare come quello turco sia un caso esemplare di un difficile equilibrio in cui la comunità internazionale, *in primis* la spesse volte ondivaga Europa, deve affrontare una grande sfida. Ritengo che tutti noi siamo consapevoli dell'importanza della Turchia, che é al tempo stesso membro della NATO, ma anche grande *player* della scena mediorientale; parte di fatto del conflitto in Siria, ma anche della questione israelo-palestinese; *partner* economico dell'Europa, ma anche protagonista di una nuova intesa, che tocca pure il tema strategico dell'energia, con la Russia.

che si presenta, per l'appunto, molto complesso. Non possiamo che osservare, con grande e giustificata preoccupazione, come fa nella sua relazione, signor Ministro, la svolta di tipo autoritario di cui è protagonista il Governo turco. turco. Non possiamo, però, permetterci, come italiani e come europei, di perdere la Turchia nel decisivo e storico ruolo di alleato atlantico e di *partner* economico. Spesso ho sostenuto posizioni critiche sulle politiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato l'azione internazionale degli Stati Uniti, dalle vicende mediorientali e nordafricane al rapporto con la Russia. Mi sembra che, anche con riguardo alla Turchia, da parte americana siano stati compiuti errori e ci siano state superficialità. Mi auguro che, al contrario di quanto già avvenuto in Nord Africa e in Medio Oriente, l'Europa abbia la forza e la capacità di una posizione propria e autonoma, che le dia un ruolo internazionale. Penso che ciò debba avvenire in primo luogo avendo il coraggio di dire chiaramente cosa si intende fare rispetto a un tema su cui, ormai da tempo immemore, da parte dell'Unione europea, ma anche della stessa Turchia, vi sono ambiguità ed esitazioni, e mi riferisco al Se si ritiene che sia interesse dell'Europa avere la Turchia tra i suoi Stati membri, si abbia il coraggio di dirlo apertamente e di comportarsi in modo coerente. Se invece così non deve essere, lo si dica in modo altrettanto aperto, avendo la capacità di lavorare per un rapporto un rapporto chiaro e corretto con la Turchia. Questa ambiguità, oggi esistente, con gravi ripercussioni, rappresenta un elemento nel quale, invece, eventuali pulsioni autoritarie e spinte antieuropee possono trovare alimentazione, come purtroppo sta avvenendo. Due anni fa, in veste di relatore della legge di ratifica dell'Accordo tra Italia e Turchia sulla giustizia, ho affermato l'utilità di tutte le forme di collaborazione con la Turchia, anche nella prospettiva di una sua eventuale adesione all'Unione europea, che è stato e costituisce un elemento fondante della politica estera italiana, in una prospettiva di contenimento del terrorismo islamico. Oggi, Oggi, con il mio Gruppo, condanno con fermezza i comportamenti che ledono la libertà di espressione, che non rispettano i diritti umani e che portano instabilità politica. Molto di quello che sta avvenendo in Turchia non ci piace, come europei e come italiani,

In questo quadro di espansione del radicalismo islamico, i cui primi segnali si sono concretizzati nei sanguinosi attentati avvenuti in Turchia, dobbiamo essere capaci di lavorare insieme all'interno dell'Unione europea per far comprendere che la preoccupazione per quanto avviene in Turchia, compresa l'ondata di arresti dopo il mancato golpe di luglio, non è una sterile ingerenza diplomatica nelle vicende interne turche, bensì una chiara posizione politica. Signor Ministro, il Gruppo AL-A dopo il suo intervento non può che condividere la posizione del Governo da lei espressa anche nel Consiglio Affari esteri dell'Unione europea del 14 novembre: mantenere le aperture alla Turchia; esigere chiarezza sul processo di di adesione turca all'Unione europea; valutare in che modo possa essere migliorato l'accordo tra Unione europea e Turchia sull'immigrazione; approfondire il tema molto importante della liberalizzazione del regime dei visti europei per i cittadini della Turchia, sostenendo il messaggio fondamentale che l'importanza di questi accordi non può far chiudere gli occhi alla comunità internazionale, all'Unione europea e all'Italia sui gravi fatti della recente scena politica turca, non ultima l'annunciata possibile introduzione della pena di morte. Su questa linea, il Gruppo AL-A garantisce la propria volontà di contribuire al formarsi e all'affermarsi di una posizione italiana sempre più forte in ambito europeo. repressive poste in atto dal presidente Erdogan dal tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016 delineano un grave mutamento del sistema politico e istituzionale della Turchia. Sono state soppresse le regole dello Stato di diritto in netta controtendenza con i principi e la strategia della modernizzazione del Paese, storicamente affidati a una visione laica e occidentale della Repubblica turca. La Turchia è attualmente un Paese nel quale la Costituzione è di fatto sospesa. Dopo il 15 luglio 2016 sono stati adottati provvedimenti repressivi nei confronti di ogni soggetto e forma di opposizione, con sistematica violazione dei diritti umani. Erdogan ha minacciato la reintroduzione della pena di morte, ha fatto arrestare i parlamentari dei partiti di opposizione e, in primo luogo, del partito HDP; perseguita i giornalisti indipendenti e gli intellettuali e ha fatto chiudere gli spazi informativi e di dialogo su Internet. Tali azioni segnano il passaggio dal presidenzialismo a un vero e proprio regime autoritario. Siamo da tempo di fronte a una sorta di guerra civile, accentuata anche dalle politiche repressive di Ezdagan in primo luogo nei confronti della minoranza curda e, più in generale, rivolte contro ogni possibile La crisi dei flussi migratori e il ruolo geopolitico della Turchia, anziché essere degli anticorpi strutturali a una deriva nazionalista, hanno rafforzato il revisionismo politico e ideologico del presidente-califfo Erdogan. Certo, l'Europa ha le proprie responsabilità nella impostazione e nella gestione di un negoziato per l'adesione della Turchia all'Unione europea, le cui contraddizioni e reciproche ipocrisie sono senz'altro una concausa perché si è determinata la situazione attuale. Inoltre, il rifiuto egoistico-nazionalista dei Paesi dell'Est europeo a una politica integrata sugli immigrati ha rafforzato oltre misura il potere contrattuale del regime di Erdogan, che utilizza i tre milioni di rifugiati presenti sul territorio come arma di ricatto nei confronti dell'Unione europea. Chiede con forza l'eliminazione del visto per i cittadini turchi entro il 2016, benché la sua *leadership* islamista rifiuta l'adeguamento della Turchia agli *standard* europei. Persegue ultimamente il sogno anacronistico della Grande Turchia minacciando di annettere territori degli Stati confinanti. Condividiamo, quindi, le posizioni assunte dal Governo italiano e ribadite oggi dal ministro degli affari esteri Gentiloni; posizioni ispirate a princìpi di cautela e di responsabilità, che devono inevitabilmente qualificare il confronto europeo e la politica estera dell'Unione europea. L'Unione europea, come richiesto dall'Italia, deve ritrovare finalmente la coesione interna per poter esercitare una seria e credibile capacità di pressione affinché vengano rispettati i diritti fondamentali in Turchia, inclusi quelli delle minoranze linguistiche. L'isolamento definitivo della Turchia è sicuramente la via sbagliata. Ma sui valori fondamentali e sui principi fondanti dell'Europa non si transige e tanto meno si concedono sconti. e tutti noi dobbiamo essere solidali con le vittime delle epurazioni e degli arresti di massa operati da Erdogan, in particolare con i nostri colleghi parlamentari Grazie

ormai da diversi mesi non passa giorno senza che dalla Turchia arrivino notizie drammatiche di arresti, di sistematiche violazioni dei diritti umani e di colpi sempre più duri alle libertà democratiche.

Davvero non è più il momento di allarmarsi: è il momento di fare delle cose, di prendere posizioni coraggiose e anche di dimostrare una volta per tutte che le parole sulla difesa dei valori europei non sono soltanto chiacchiere. Signor Ministro, noi siamo molto convinti del fatto che la repressione in atto in Turchia e la edificazione di un vero e proprio sostanziale sostanziale regime dittatoriale non siano iniziate semplicemente nella notte tra il 15 e il 16 luglio scorsi, quella del tentativo di colpo di Stato: la marea di arresti, le tantissime espulsioni dalla pubblica amministrazione, l'abolizione dell'immunità parlamentare e la censura sull'informazione che si è scatenata dopo il tentato *golpe* - e che peraltro non accenna a placarsi erano ampiamente annunciate e anticipate da uno stillicidio di misure liberticide che già da tempo era cominciato. Due anni fa Erdogan replicò alla richiesta di chiarimenti europei sull'arresto di 27 giornalisti dissidenti dicendo, testualmente, che l'Europa deve farsi i fatti propri. Noi crediamo che il problema sia stato proprio il fatto che l'Europa scelse allora,

pur sapendo che questo equivaleva a una vera e propria mano libera lasciata al dittatore turco. E purtroppo l'Europa continua a chiudere gli occhi ancora adesso. Erdogan serve a contenere l'ondata migratoria e, allora, cosa volete che siano migliaia di arresti di fronte a un fatto come questo? Forse i princìpi valgono fino a quando non intaccano gli interessi concreti

che, a suo parere, i negoziati per l'ingresso della Turchia nell'Unione europea non debbono essere interrotti e che la decisione sull'avvicinarsi o meno all'Europa deve essere presa non in Europa, ma in Turchia.

La Turchia di Erdogan, purtroppo, ha già preso la sua decisione e la conferma ogni giorno. La prende quando arresta, senza motivo e senza garanzia, Demirtaș e la *leadership* dell'HDP, partito al quale, da parte del nostro Gruppo e del nostro partito, vanno la più totale solidarietà e il più totale sostegno,

Ora è l'Europa che deve prendere delle decisioni. Innanzitutto, deve prendere una decisione su un punto di fondo: se vuole difendere o meno i propri principi.

se necessario anche pagandone il prezzo. Ciò vuol dire, per l'appunto, dimostrare che l'Europa considera quello che sta accadendo in Turchia non più tollerabile. Se invece, in base a una davvero miope *Realpolitik*, dovessimo scegliere di tradire questi principi, pagheremmo un prezzo salatissimo, perché nessuna grande democrazia può sopravvivere a lungo fondandosi sul rinnegamento della propria civiltà e della propria ragione d'essere. Noi pensiamo che l'Italia debba muoversi in maniera molto forte in questa direzione, e più forte rispetto a quanto ha fatto finora, fino a immaginare misure drastiche, anche ritirando l'ambasciatore, se occorre, e anche chiedendo la sospensione dei trattati internazionali, se occorre. Deve muoversi subito e deve muoversi anche in autonomia. Noi pensiamo che non sia più una questione che possiamo trattare come una delle tante cose che accade nel mondo. No: la solidarietà nostra a Demirtaș, alla *leadership* dell'HDP, ai militanti curdi che sono stati in questi mesi anche oggetto di drammatici attentati, la vogliamo ribadire oggi con tutta la forza che abbiamo Cari colleghi, cinque minuti per parlare di un problema come quello della Turchia e della vicenda che quel Paese sta vivendo - voi capite - sono un po' pochi.

il detto perché abbiamo sentito la sua condanna in ordine ai parlamentari privati della loro libertà; ma anche il non detto, o il sottinteso, o l'accennato, perché l'Europa deve farsi un serio esame di coscienza sulle inadeguatezze, incapacità previsionali e omissioni che ha avuto in tempi non sospetti nei confronti della Turchia. Se oggi la Turchia sta cavalcando una sorta di visione neo-ottomana, forse è anche per chi gli ha chiuso le porte nel 2003 - parlo di Schröder e Chirac mentre alcuni Paesi come l'Italia - allora c'era il Governo Berlusconi, ma successivamente Prodi ha tenuto la stessa linea avevano in qualche modo cercato di tenere aperto a questo grande Paese, fondamentale per gli equilibri dell'Europa e del Mediterraneo, le proprie porte. porte. Caro collega De Cristofaro, capisco la sua indignazione e la comprendo fino in fondo, ma dico ai colleghi parlamentari di attenzione: noi non possiamo chiudere le porte dell'Europa e dell'Italia alla Turchia e, pur in presenza di visioni diverse con quel Paese o di opinioni diverse tra i Governi o di opinioni diverse tra i Parlamenti - io stesso ho parlato con il mio collega Presidente della Commissione esteri nei giorni scorsi - dobbiamo sforzarci di tenere aperto il dialogo. Sarebbe un errore storico mortale per l'Europa e il Mediterraneo se sospingessimo la Turchia su una deriva da cui potremmo avere solo danni enormi. Cari colleghi, vorrei dirvi una cosa. Ho piacere di tutta l'indignazione che c'è e in parte la condivido, ma la notte del *golpe* in Turchia ho aspettato troppo tempo per vedere la stessa indignazione nell'esprimere solidarietà a Erdogan, che in quel momento era il il soggetto passivo di ciò che si stava perpetrando. Quel silenzio è stato troppo lungo. Quella esitazione, anche degli europei, è stata troppo lunga e su questo dobbiamo avere le idee chiare. tempo, va approfondita la cosiddetta pista gulenista, che mi sembra sia stata troppo superficialmente scartata anche dai mezzi di comunicazione di massa del nostro Paese. Che scuole coraniche

ideologizzato in gran parte degli apparati statali di quel Paese è una realtà incontestabile. Credo che oggi noi dobbiamo metterci nei panni di chi ha subito un *golpe*, di chi subisce costantemente attentati terroristici e di chi riceve sul proprio territorio milioni di rifugiati, molti dei quali sono lì altrimenti starebbero qui. Con tutti i limiti giustamente ricordati dal ministro Gentiloni, quell'accordo,

Signor Presidente, tutto quello che sta avvenendo in Turchia in questi mesi noi del Movimento 5 Stelle, che non siamo certo dei profeti, lo avevamo previsto già lo scorso anno, in occasione del tragico attentato del 10 ottobre contro un corteo pacifista ad Ankara. Eppure nello stesso periodo, quando era ormai chiaro il legame tra il Governo turco e le milizie islamiche che in Occidente si definiscono moderate, ci si sarebbe dovuti aspettare che la Turchia voleva qualcosa di più che appoggiare acriticamente l'Occidente nella crociata contro Assad. Erdogan poggia le sue basi sull'Islam e sul fortissimo sentimento nazionalista. La maggioranza dei suoi cittadini non nutre alcuna simpatia per le nostre forme politiche, ma - anzi - le percepisce come una minaccia all'indipendenza del Paese, vedendo nel Presidente turco un padre della Patria e non un sanguinario dittatore. Cosa avrebbe dovuto fare l'Unione europea? Partiamo da quello che non avrebbe dovuto fare per non risultare poco credibile. Partiamo dai fondi dell'Unione europea concessi alla Turchia. Dei soldi corrisposti dall'Unione europea, una volta attraversato il Bosforo, non c'è traccia: manca la trasparenza su come le autorità turche utilizzino i fondi dei cittadini europei. E di soldi ne abbiamo dati, eccome. Nell'arco degli ultimi diciotto anni abbiamo versato - o siamo in procinto di farlo - quasi 40 miliardi di euro attraverso le linee di finanziamento, i fondi di preadesione e l'accordo sui migranti. Se avessimo subordinato la concessione dei fondi alla pretesa di trasparenza ed efficienza, oggi dovremmo avere contezza di ogni centesimo speso, mentre non sappiamo, se non a grandi linee, che fine hanno fatto tutti quei soldi. Sono stati forse usati, almeno in parte, per rimpinguare le forze di sicurezza turche e finanziare le milizie islamiche in Siria? Eccoci dunque alla seconda contraddizione: rimanere silenti di fronte alle innumerevoli violazioni delle regole democratiche e dei diritti umani. Di momenti bui la democrazia turca ne ha conosciuti a bizzeffe, soprattutto negli ultimi due anni quando, tra attentati e la fine della tregua con il PKK, i turchi sono stati messi all'angolo - almeno questa è la loro impressione - fino a quando l'*establishment* che governa la cosiddetta comunità internazionale ha deciso di fare fuori Erdogan con il tentativo di colpo di Stato, che non poteva avere successo - e, infatti, non l'ha avuto - permettendogli di puntellare il suo potere e passare all'attacco. Pochi ormai sono i dubbi che quel tentativo non fosse ispirato da qualcuno in Occidente, visto che tutto è partito dalla base militare NATO di Incirlik. Dei turchi possiamo dire tutto, ma sono sicuramente più complottisti della Clinton, che vede *hacker* russi ovunque, e quindi hanno mangiato la foglia. Da lì a poco la riapertura delle relazioni con Putin, messaggio forte e chiaro soprattutto alla casta politica europea e statunitense. Altro che lezioni di politica estera! è anche dell'inetta casta europea che, a forza di pragmatismo e affarismo di bassa lega, se n'è fregata della prospettiva e ha guardato solo alla contingenza. I tempi della storia non sempre collimano con i desideri. È successo a Hitler, che pensava di conquistare la Russia stalinista in pochi mesi; è successo all'asse USA-UE, che pensava di far fuori Assad con la stessa celerità con cui aveva assassinato Gheddafi. Il prolungarsi della guerra ha costretto gli americani ad armare i curdi, destabilizzando di conseguenza anche la Turchia. Allora cosa consigliano di fare i 5 Stelle? Anzitutto, allo stato attuale non è possibile continuare ad appoggiare un ingresso della Turchia nell'Unione europea per almeno due motivi: il primo è che la Turchia non ha nulla di democratico, almeno nel senso in cui noi europei intendiamo la democrazia, seppur tra mille contraddizioni. Il secondo motivo è che liberalizzare i visti dei cittadini turchi, e quindi abbassare i controlli alle frontiere, ci porrebbe di fronte ad un rischio attentati. L'unica strada per evitare di rimanere ostaggio di Erdogan è la risoluzione del conflitto siriano. Poi si sa, signor Presidente, signor Ministro, noi 5 Stelle siamo populisti, gli esperti di politica estera siete voi. Ma, per come stanno andando le cose, dubito fortemente che riuscirete a risolvere questi problemi e in ogni caso, nell'interesse di tutti i cittadini europei, vi faccio i miei migliori auguri per il futuro, anche se, da quello che vedo, non vi è rimasto più molto tempo. *(Applausi

Da tempo la Turchia ha intrapreso un percorso di adesione all'Unione europea che l'Italia, forse più di altri, ha assecondato, con un amplio schieramento politico. Da parte sua, Ankara è sempre stata consapevole che tale percorso aveva e ha delle regole da rispettare. Oggi, tuttavia, la situazione in quel Paese è sempre più difficile, in un crescendo di azioni e iniziative culminate con l'arresto dei *leader* del secondo partito di opposizione - come ha ben ricordato il Ministro da parte del Governo in carica, difficilmente compatibili con le suddette regole dell'Unione europea. Non v'è dubbio che oggi la Turchia costituisca un elemento di grande preoccupazione e delicatezza. pur comprendendo gli interessi geopolitici ed economici che ci legano a quel Paese, crediamo che l'Europa, ma anche l'Italia e questo Governo, non possano barattare la collaborazione sul fronte migratorio col silenzio sulle ansie e sulle inquietudini che l'operato del Governo turco ha scaricato su uno scenario internazionale già gravido di pericolose tensioni. Lo Stato turco ha contribuito nell'ultimo periodo a turbare consolidati equilibri regionali e non è del tutto esente dal caos che è di fronte ai nostri occhi, mentre tenta di estendere la sua influenza nell'area mediterranea e nel Corno d'Africa, dove per primi hanno riaperto l'ambasciata a Mogadiscio. L'iniziale espansione del cosiddetto califfato ha goduto del flusso in territorio turco di migliaia di jihadisti, transitati in entrata e in uscita dal fronte, tra i silenzi delle evanescenti e superficiali cancellerie occidentali. Il Paese, certo, ha subito anche attentati devastanti che hanno mietuto vittime innocenti, per cui abbiamo manifestato la dovuta solidarietà. Ma la situazione, Ministro, è sempre più complessa e avrebbe dovuto imporre anche al nostro Paese una valutazione dettagliata delle possibili conseguenze di ogni decisione da assumere, compresi i tre miliardi di euro dati dall'Unione europea alla Turchia per frenare il flusso di profughi, nel mentre si continua a turlupinare il nostro Paese sulle quote di migranti da ricollocare. Lei, signor Ministro, si è dichiarato contento per aver trovato comprensione e incoraggiamento da parte delle istituzioni europee nelle scorse ore per l'iniziativa italiana in relazione agli accordi con alcuni Paesi africani. Nel frattempo continuiamo a importare clandestini a migliaia al giorno, con le nostre navi a ridosso delle coste libiche; vediamo da vicino barche, gommoni e scafisti, ma non si interviene in quei porti, preferendo mandare centinaia di paracadutisti a Misurata. Tutto ciò accade a causa di una politica estera sempre più deficitaria, con un Governo che, al di là di vuoti *slogan*, ha poca credibilità internazionale, sempre più al traino degli Stati Uniti del presidente Obama, con cui con cui siamo stati alleati e sempre allineati alla sua disastrosa politica estera che ha messo a rischio il mondo, anche a causa di un Ministro degli esteri che, per fortuna, non è divenuta Presidente degli Stati Uniti. È una politica estera, quella italiana, che si trascina stancamente tra *gaffe* e propaganda, provincialismo e mancanza di autonomia. In Libia abbiamo sponsorizzato un Governo fantoccio, che a otto mesi dall'insediamento è ben lungi dall'unificare il Paese, ma - ciò che è peggio - non è riuscito a fermare un solo barcone col suo carico di disperati. È una situazione che vi rende complici morali degli scafisti. scafisti. Non si comprende, poi, Ministro, quale sia l'utilità di aver sostenuto un Governo che, in un punto del suo programma, prevede che l'unica fonte del diritto sarà la *sharia* - una domanda che io stesso le ho posto in Commissione, ma alla quale lei non ha risposto

Nel frattempo, ci siamo anche allontanati dall'Egitto, al quale, con pressappochismo e superficialità, il Governo italiano ha negato, dopo il ritiro dell'ambasciatore per il caso Regeni, i pezzi di ricambio degli aerei F-16. Un atto ostile nei confronti del nostro principale alleato in Nord Africa, di cui il nostro Paese è il secondo *partner* commerciale. In un momento caotico che vede il Mediterraneo incendiarsi, le relazioni con la Turchia non offrono le certezze di un tempo, e sarebbe opportuno insistere con quel Paese per affermare senza impaccio e timidezza i principi e i valori della democrazia che, con molta fatica, ancora si perseguono nella cara, vecchia Europa. Presidente - e concludo - che il nuovo Presidente degli Stati Uniti ponga serio rimedio a quell'era oscura del duo Obama-Clinton, che dall'avallo alle rovinose primavere arabe alle valutazioni errate sui presunti ribelli anti Assad in Siria, sino alle scellerate e inutili sanzioni alla Russia, hanno messo a rischio l'intero l'intero Pianeta: altro che *global warming*! L'augurio è che possa quanto prima avviarsi una stagione in cui si attenuino le tensioni tra Stati Uniti e Federazione Russa e si avvii un proficuo negoziato in cui inserire le relazioni turco-europee, sperando di definire quindi un costruttivo rapporto che soddisfi anche i nostri interessi geopolitici. *(Applausi

complesso, che cinque minuti di intervento francamente non consentono di esaminare compiutamente. Essere equilibrati vuol dire, intanto, ricordare che la Turchia è un grandissimo Paese, che ha di sé l'idea di essere una grande potenza e che nel corso di questi ultimi anni, per la verità, con la Presidenza di Erdogan, ha accresciuto sia la sua dimensione, sia il suo interventismo nella politica internazionale.

Siamo di fronte a un Paese che ha una storia lunga, che viene, come veniva ricordato nel dibattito, da Sèvres, dal trattato di Losanna, dal fatto che quel Paese ha trovato i propri confini e la propria identità dopo la sconfitta della guerra del 1915-1918 e dopo l'annullamento dell'Impero ottomano. È un Paese che ha cercato negli anni, continuamente, soprattutto nel periodo di Ataturk, di ritrovare la propria dignità nazionale, la propria forza, la propria

più di un'ipotesi. Erdogan coltiva un'ipotesi da grande P2 ramificata in tutta la struttura dello Stato: nella polizia, nelle Forze armate, nell'università, nei giornali, cioè in tutte quelle strutture che nel corso di questi mesi ha epurato con centinaia di migliaia di licenziamenti e con decine di migliaia di arresti.

che ha tolto le guarentigie parlamentari e la protezione alla politica dei parlamentari -, è arrivato ad arrestare i parlamentari dell'HDP, partito cui il Partito Democratico rivolge la propria solidarietà e il proprio sostegno, sapendo che è l'unico partito, come lei ci diceva,

Ma da qui ad andare oltre, cioè a dire che dobbiamo inasprire i nostri rapporti nei confronti della Turchia,

perché quando si lascia qualcuno a bagnomaria per molto tempo, senza dargli la possibilità reale di entrare nel novero delle Nazioni europee, poi finisce che salta dall'altra parte, in Europa non viene più e combina guai peggiori. Noi crediamo di avere un dovere. Siamo un grande Paese democratico un grande Paese democratico e come tale abbiamo il dovere di aiutare la Turchia a uscire da una fase certamente difficile, inducendo Erdogan a non compiere scelte ancora più scellerate di quelle che ha fatto, ma contemporaneamente mantenendo aperti tutti quei margini di relazione e di trattativa che ci consentano di rivedere la Turchia come un Paese fondamentale in quello scacchiere. Lo dico tanto più adesso che gli Stati Uniti d'America appaiono orientati su quello scacchiere verso la Russia e probabilmente anche verso il rapporto con la Turchia, sapendo che anche l'Italia lì può giocare un ruolo molto importante, proprio perché noi non abbiamo lasciato la Turchia fuori dall'Europa volendocela lasciare e abbiamo una lunga tradizione tendente, al di là di ogni altra cosa, a cercare di portare questo Paese dentro l'Unione europea. Se l'avessimo fatto, se l'avessimo almeno messa in una situazione allargata, probabilmente oggi avremmo tutti molta meno difficoltà ad affrontare una situazione di questo genere e non avremmo abbandonato la Turchia al suo destino. Questa è l'unica cosa che non dobbiamo fare:

colleghi, con la morte, lo scorso 8 novembre, di Umberto Veronesi scompare non solo un oncologo di fama mondiale, ma anche un illustre studioso e un uomo delle istituzioni, servite come Ministro della sanità tra il 2000 e il 2001 e come senatore nella scorsa legislatura. Umberto Veronesi nasce nella periferia di Milano il 28 novembre del 1925. Dopo aver conseguito, all'inizio degli anni Cinquanta, la laurea in medicina e chirurgia, si specializza nello studio e nella cura delle patologie tumorali. Dopo alcune esperienze professionali in Gran Bretagna e Francia, inizia la collaborazione come volontario presso l'Istituto nazionale dei tumori, di cui diviene direttore generale nel 1975. Nel 1965 contribuisce alla nascita dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e alla fondazione, nel 1982, della Scuola europea di oncologia. Dal 1985 al 1988 presiede l'Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro. Nel 1991 fonda l'Istituto europeo di oncologia, polo di ricerca di avanguardia del settore, di cui è direttore scientifico dal 1994 al 2000 e, successivamente, dal 2001 al 2014. Nel 1993 viene nominato membro della commissione nazionale incaricata di predisporre un piano contro le malattie tumorali e dal 2003 promuove l'attività della Fondazione a lui intitolata, che ha portato vasti contributi al progresso scientifico e alla ricerca nel settore dell'oncologia, della cardiologia e delle neuroscienze. Tra le iniziative della Fondazione, si ricorda in particolare il progetto Science for peace, avviato nel 2009 sostenuto da un movimento internazionale per la pace guidato da illustri scienziati, tra cui diversi premi Nobel, con lo scopo di affrontare con rigore scientifico le cause alla base di conflitti e disuguaglianze, promuovendo strategie concrete per il loro superamento. Dal 2010 presiede il comitato scientifico della Fondazione Italia-Stati Uniti. Nella veste di Ministro della sanità nel secondo Governo Amato, si impegna per l'introduzione di una normativa sul divieto di fumo nei luoghi pubblici, ponendo così le basi per l'entrata in vigore nel 2003 della cosiddetta legge Sirchia. Altresì, sempre in tale veste, introduce la gratuità di forme di *screening* preventivo di patologie tumorali. Eletto al Senato nelle liste del Partito Democratico in occasione delle consultazioni del 2008, entra a far parte della Commissione istruzione e mette la sua competenza ed esperienza al servizio del del legislatore, impegnandosi in particolare sulle tematiche connesse alla ricerca scientifica, nonché per l'introduzione di una normativa sulla disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel febbraio del 2011 si dimette dal senatore per ricoprire l'incarico di presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, carica che abbandona nel settembre del medesimo anno, a seguito dell'esito del *referendum* contrario alla produzione in Italia di energia elettrica di origine nucleare. Il nome e la memoria di Umberto Veronesi resteranno legati principalmente al prezioso contributo fornito per la prevenzione e la cura del tumore al seno, con particolare riferimento all'invenzione della chirurgia conservativa e all'utilizzo di tecniche innovative in grado di limitare l'impatto psicologico ed estetico della malattia, oltre che naturalmente di aumentare le possibilità di completa guarigione. sua attività di medico ha contribuito alla salvezza di tante vite umane, coniugando costantemente la competenza professionale a un tratto inconfondibile di affabilità e garbo umano. Unanimemente riconosciuta la sua capacità di entrare in empatia con il paziente. Nel corso della sua lunga vita Umberto Veronesi ha preso parte in prima persona anche ad iniziative numerose di impegno civile, senza mai rinunciare ad assumere posizioni chiare su tematiche controverse e dibattute. Tra queste, le iniziative sulla legalizzazione delle droghe leggere e sul relativo utilizzo a scopi terapeutici, l'approccio scientifico agli organismi geneticamente modificati, la promozione dell'alimentazione vegetariana e la difesa degli animali, la possibilità di ricorrere al testamento biologico evitando forme di accanimento terapeutico e il sostegno all'utilizzo dell'energia nucleare. Il contributo intellettuale e l'ampia produzione saggistica di Veronesi, che hanno contribuito ad avvicinare larghi settori dell'opinione pubblica a tematiche scientifiche, sono stati sempre orientati a favorire un approccio razionale alla ricerca, avulso da preconcetti ideologici, in linea con la sua formazione di scienziato laico. «Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza e ragione»: è, per certi versi, la sintesi del suo lascito intellettuale, raccolto dall'omonima Fondazione. È il messaggio dell'uomo Veronesi, ma anche dello scienziato che, rivolgendosi ai giovani medici e ricercatori, scriveva: «Siate dubbiosi, siate trasgressivi, se trasgredire significa andare oltre il limite del dogma o la rigidità della regola», a dimostrazione di quella curiosità intellettuale e di quell'amore per la ricerca che hanno rappresentato i tratti ispiratori della sua azione di medico, di studioso, di uomo delle istituzioni. Saluto il figlio Alberto, presente in tribuna, al quale rinnovo l'espressione di profondo cordoglio e partecipazione, e invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.

Presidente, per i senatori del Partito Democratico Umberto Veronesi non è stato solo un grande medico e un grande scienziato, perché nella precedente legislatura è stato un senatore del nostro Gruppo e un amico prezioso. Ed è con questo spirito di amicizia che tutti noi oggi salutiamo il figlio Alberto, Grazie Con Umberto Veronesi siamo stati seduti negli stessi banchi di Palazzo Madama e abbiamo condiviso le stesse posizioni parlamentari. In quegli anni, ciascuno di noi gli si

Umberto Veronesi rispondeva con generosità e con quel tratto umano che chi lo ha conosciuto ben ricorda. Per noi è stato un collega molto importante, che ha dato autorevolezza al nostro Gruppo non solo con la sua scienza, ma anche per le parole straordinariamente semplici con cui sapeva mostrare il suo punto di vista su questioni molto delicate e, oggi pomeriggio, il tempo di cui disponiamo non è sufficiente a rendergli l'onore che merita e per esprimergli tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza. Presto le senatrici e i senatori del Partito Democratico promuoveranno in suo onore una giornata di studio e di riflessione, così da poterlo ricordare

l'indipendenza della ricerca e del metodo scientifici, il testamento biologico per il quale si è tanto battuto ed anche quel difficile ma necessario rapporto tra scienza e politica che, da Ministro della salute e da senatore, Umberto Veronesi ha sempre inteso non come confronto tra due poteri, ma come servizio al suo Paese. Lo abbiamo conosciuto nella dimensione molto particolare delle Aule parlamentari, dove spesso la politica nasconde la vera natura di ciascuno di noi. Umberto Veronesi era sempre lo stesso, in Senato o in ospedale, con gli amici o con chi incontrava per caso e a tutti mostrava con trasparenza le sue passioni, le sue attenzioni e le sue curiosità. Era un uomo aperto alla vita, una personalità ricca di interessi, nutrita da una vastissima esperienza culturale, professionale e scientifica. Il tutto tenuto insieme da una grande passione per una missione pubblica molto intensa, chiara a chiunque abbia avuto la fortuna di condividere con lui le grandi battaglie civili per le quali si è battuto. Per Veronesi ogni paziente era, prima di tutto, una persona. Una persona che, sia che l'avesse in cura, sia se per caso gli veniva richiesto un consiglio, era sempre il centro assoluto della sua attenzione.

dei risultati scientifici delle sue ricerche e dei progressi che raggiungeva con una esperienza quotidiana che ha praticato fino alla fine. Tutti sappiamo quanto l'umanità gli sia in debito per i risultati straordinari raggiunti nella cura e nella prevenzione del cancro. E sappiamo quanto le donne, in particolare, debbano alla genialità con la quale le ha sempre curate, proteggendone la dignità e la femminilità. Aveva la vista lunga e mi ha colpito sapere che sognasse di riuscire a vedere, prima di morire, la vittoria definitiva della scienza sul cancro. Il suo era un desiderio grandioso e, nonostante i grandi progressi cui lui stesso ha così tanto contribuito, non lo ha visto completamente realizzato nel lungo tempo della sua vita. Ma noi sappiamo che quando l'uomo potrà dire di aver definitivamente battuto il cancro, il merito principale sarà di Umberto Veronesi, grande italiano e grande milanese.

Umberto Veronesi è stato una grande e bella persona. Uno scienziato eccellente, per molti anni all'avanguardia sul piano internazionale. Grande organizzatore, sapeva che la sola scienza non era sufficiente ed è stato in grado sempre di mettere assieme un *team* di persone in grado di assecondarlo e di aiutarlo, a beneficio del paziente. È stato capace di trovare finanziamenti privati cospicui, sempre ad esclusivo beneficio del paziente. È stato un comunicatore capace ed è stato in grado di far capire all'opinione pubblica e all'interlocutore profano in materia medico-scientifica come vanno affrontati determinati problemi complessi e dolorosi. Soprattutto, aveva una straordinaria disponibilità umana. In ogni giorno della sua lunghissima attività professionale, Umberto Veronesi si è posto con tutti i suoi pazienti come una persona che partecipava al dolore fisico e alle tensioni psicologiche di donne e uomini, che trovavano in lui un sostegno vero e partecipato. È stato un uomo libero e sincero. Ha sempre sostenuto i suoi convincimenti con onestà intellettuale, rispettando le idee diverse dalle sue, senza inseguire la popolarità a tutti i costi. In libri e interviste ha fatto considerazioni che ci hanno fatto pensare su aspetti importanti della vita. Grazie a donne e uomini come Umberto Veronesi, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, l'età media è sensibilmente cresciuta e la qualità della vita della terza, della quarta e della quinta età è sensibilmente migliorata. Forza Italia lo saluta e gli rende omaggio con commozione ed affetto e partecipa al dolore del figlio Alberto con vera commozione

il nome di Veronesi è legato a grandi contributi scientifici e culturali, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, per i quali è stato insignito con dieci lauree *honoris causa* in medicina, riconosciutegli dall'Argentina al Brasile, dalla Grecia alla Spagna. La sua vita, di fatto, è stata spesa nell'attività clinica e di ricerca sulla prevenzione e sulla cura del cancro in generale. Ha fondato l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), la Scuola europea di oncologia e l'Istituto europeo di oncologia. Le sue parole d'ordine erano ricerca e laicità: ricerca pubblica, libera dagli interessi dei grandi gruppi farmaceutici. Tra i grandi lasciti e le conquiste che dobbiamo a Veronesi, tra gli altri, voglio sottolineare in modo particolare i risultati conseguiti nelle ricerche sul linfonodo sentinella, campanello sullo stato di avanzamento della malattia oncologica del seno, e la terapia adiuvante, un tempo osteggiata da quei medici che non amavano lavorare in *equipe*. ha infatti voluto mettere il paziente al centro e la medicina al suo servizio. In particolare, le donne devono molto alla figura dell'oncologo milanese, per la dimensione e la diffusione della chirurgia conservativa per alcuni tipi di tumori mammari. I dati preliminari degli studi in tali ambiti vennero pubblicati nel 1981, sul prestigioso «New England journal of medicine» e da quel momento ebbe inizio nel mondo la grande evoluzione di pensiero che permise, negli anni successivi, alle donne con tumore al seno di evitare l'asportazione della mammella con la quadrantectomia abbinata alla radioterapia, a minor impatto psicologico, estetico e sessuale. Più recentemente le sue ricerche sono proseguite sulla stessa strada, con la biopsia del linfonodo sentinella, per evitare la dissezione ascellare nei casi in cui i linfonodi siano sani. In questi ultimissimi anni ha rivoluzionato le procedure della radioterapia dei tumori mammari, introducendo la radioterapia intraoperatoria, che si esaurisce in una sola seduta, durante l'intervento stesso. Ovviamente c'è ancora molto da fare nell'ambito del tumore al seno, bisogna estendere la fascia di età in cui viene effettuato lo *screening* mammografico a tutte le donne, dall'età di 40 anni in poi. Tutto ciò per far sì che

medicina e fare ricerca dove è possibile. Si cura meglio dove si fa ricerca e quindi occorre prevedere forti incentivazioni per chi investe in ricerca e lo fa seriamente, in modo tale che il lascito umano, scientifico ed etico di Umberto Veronesi non si disperda inutilmente, ma possa essere a maggior ragione concime per le future ricerche e innovazioni in campo oncologico. Signor Presidente, è stato detto molto di Umberto Veronesi, molte cose belle, soprattutto sui suoi grandi meriti di medico e certamente Veronesi è stato un grande oncologo e un grande scienziato. Ma Veronesi è stato molto di più: è stato, innanzitutto, un grande uomo che ha profondamente amato la vita e che ha cercato, con le sue conoscenze, le sue scoperte, la sua sensibilità e la sua passione, di insegnare a tutti noi ad amare la vita,

Veronesi amava la vita tutta e aveva grande rispetto degli esseri viventi tutti, inclusi gli animali, e questa era una delle ragioni della sua scelta di essere vegetariano. vegetariano. Il suo impegno più grande è stato combattere il male e il cancro è una delle espressioni del male. L'ha combattuto per ridare la gioia di vivere a chi la stava perdendo, ma non possiamo dimenticare le sue battaglie affinché il momento della morte fosse il più sereno possibile, quando non più rinviabile. Ha combattuto perché nel momento delicato del passaggio tra la vita e la morte non venisse calpestata la dignità umana. Ha combattuto perché venisse affermato il diritto all'autodeterminazione dell'uomo e ha combattuto perché la pietà, quella vera, superasse i limiti ideologici e religiosi. Veronesi è stato davvero un uomo molto coraggioso, forte delle sue convinzioni basate sulla logica, ma una logica supportata dalla sensibilità umana, ha affrontato con grande lucidità argomenti delicati, tabù in Italia, come quello dell'eutanasia e lo ha fatto sempre con la massima onestà intellettuale. credo - e mi appello a tutti i colleghi senatori, in questo momento - che per ricordarlo davvero, per rendere omaggio a Veronesi, dovremmo avere anche noi un po' di coraggio, anche solo una piccola parte del coraggio che ha avuto lui, e affrontare senza paura questioni importanti, a mio avviso non più rinviabili, come il fine vita.

ringraziando davvero di cuore il professor Umberto Veronesi e tutta la sua famiglia, in particolar modo il figlio Alberto qui presente. Vorrei ringraziarlo per tutto ciò che ci ha regalato e ci ha insegnato.

ho avuto anche la fortuna di capire, vedendo lui operare, pioniere della quadrantectomia e della conservazione

è stato un compagno socialista, un collega dell'assemblea nazionale del PSI. Grazie alla lungimiranza di Bettino Craxi era stato chiamato come figura professionale della scienza, poiché i socialisti hanno sempre avuto grande attenzione per la ricerca, la scienza e gli uomini che hanno fatto grande in Europa e nel mondo l'Italia e Umberto era uno di questi. Quindi, con lui ho condiviso per anni il garofano che tengo in mano,

scientificamente e poi dal punto di vista legislativo la gravità del fumo per l'insorgenza di patologie croniche, di patologie cardiovascolari e neoplastiche. è stato molto di più. È stato un grande pacifista.

Si rendeva conto che il medico ha una formazione professionale di gran lunga superiore a molte altre figure, mentre è il fanalino di coda, dal punto di vista del riconoscimento anche economico, rispetto ad altre professioni e categorie (ne voglio citare una su tutte: quella dei magistrati, che guadagnano il doppio o il triplo e non rischiano nulla, come invece i medici). Ricordiamo che ha avuto anche il coraggio di presiedere l'Agenzia per la sicurezza nucleare italiana e, quando qualcuno non gli ha dato i giusti riconoscimenti e la giusta sede, si è anche dimesso per protesta. È stato un grande scienziato e un grande politico; lo ricordo, in questo momento, soprattutto come un grande socialista che ha saputo, anche nei momenti difficili, schierarsi contro certe superstizioni, come la terapia Di Bella, che ha avuto il coraggio di denunciare, così come ha avuto il coraggio di denunciare ricerca sugli organismi geneticamente modificati era da continuare a perseguire perché possono curare le persone e quindi non si è schierato con il falso populismo contro questa forma di ricerca. Ciao, Umberto.

per la sua vita politica e per la sua vita di medico, di ricercatore, di docente, di persona impegnata nel sociale e su temi che erano e sono eticamente sensibili. A Veronesi si riconosce la grande valentia di clinico chirurgo per aver individuato tecniche diagnostiche e, ancor più, di ordine chirurgico che hanno assicurato dignità alle donne,

nella commemorazione - di una laicità di ordine contenutistico, un dibattito molto vivo, che non possiamo assolutamente cancellare in quest'Aula. cui la posizione del professor Veronesi era antropologicamente ben specifica e si richiamava ad una corrente di pensiero in ambito bioetico che si chiama «funzionalismo», dove la dignità della persona veniva riconosciuta, sì, nella sua intrinseca esistenza, ma era sicuramente una dignità che veniva condizionata dalla sua qualità di vita. Ecco per quale motivo il riconoscimento di una sinonimia tra dignità e qualità di vita lo ha portato ad essere fautore di quegli interventi in ambito bioetico e direi ancor più, in quest'Aula, di ordine biopolitico di grande interesse,

dell'uso degli embrioni per la ricerca, ma era anche fortemente fautore non tanto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, quanto delle disposizioni anticipate di trattamento e del testamento biologico. Detto in altri termini, era a favore anche di procedimenti di ordine eutanasico, sia nella forma attiva, che nella forma passiva. Si riconosce e riconosco al professor Veronesi, anche in ragione di una dialettica garbata e contenutisticamente forte, che ha caratterizzato alcuni momenti del nostro vivere, nell'ambito dei temi della bioetica e della biopolitica, una laicità ed una onestà nella sua argomentazione che lo portava ad essere testimone e non solo fautore di ordine teorico di procedure che potevano essere considerate lesive della dignità della persona. È una laicità, quindi, che veniva riconosciuta nell'ambito della sua attività attività di ricerca e non solo perché, come lui ha ripetuto molte volte, bisogna essere anche trasgressivi. Ma la trasgressione, nell'ambito della ricerca, è un fondamento, perché se non si è trasgressivi, se non si va oltre, nell'ambito della ricerca ci si ferma su posizioni assunte come forza, senza interrogarsi. Il fondamento della ricerca è interrogarsi,

terapeutico. Il nostro ricordare Veronesi è un ricordare lo scienziato, il ricercatore, il grande clinico chirurgo che ha saputo suscitare dibattiti interessantissimi e di sana provocazione intellettuale e, perché no, spirituale, nella ricerca, forse, di un percorso che non che non è comune ma ha una finalità unica, che era sempre il bene ed il benessere della singola persona, di una donna, in questo caso, affetta da patologie tumorali. Credo fermamente che l'apporto dato dal professor Veronesi sia stato, non solo significativo, ma direi unico anche per quanto riguarda l'eleganza nella relazionalità assistenziale che egli sapeva brillantemente curare,

Signor Presidente, novant'anni spesi molto bene. Si è spento a novant'anni uno dei più grandi talenti della chirurgia mondiale, Umberto Veronesi, un innovatore, colui che ha inventato tecniche chirurgiche per intervenire su donne affette da tumore al seno. Veronesi amava dire che una donna doveva uscire dalla sala operatoria così come era entrata. Quando, nel 1969, espone a Ginevra, davanti a un consesso mondiale, la sua ricerca sulla quadrantectomia (cioè l'intervento che limita l'esportazione al quadrante mammario sotto cui c'è il nodulo tumorale, tumorale, considerato non invasivo rispetto all'allora vigente dogma della mastectomia) viene ascoltato quasi con fastidio. Da lì tutta una serie di ricerche che lo porteranno a intervenire su un all'epoca, veniva considerato assolutamente non guaribile. Fermo sostenitore dell'utilità della prevenzione e attento alla psicologia del paziente, Veronesi ha promosso la diffusione di stili di vita sani e di alimentazione corretta.

perché avevo promesso a me stesso che sarei morto dopo aver visto il cancro sconfitto, e temo non succederà. Però posso dire che una battaglia importante l'ho vinta, ed è quella di convincere i miei colleghi a cambiare strategia contro i tumori». In un'intervista Veronesi dichiarava che l'ultimo tratto della sua vita era bellissimo: «Non devo più fare a pugni per fare carriera, e questa è una gran gioia. Poi si è arricchiti dalla conoscenza, dall'esperienza e da una filosofia di vita molto più distaccata e imparziale. Il metro di giudizio è più indipendente e meno passionale. Quindi è giusto vivere fino all'ultimo giorno senza il desidero di andarsene, però è anche giusto accettare la morte come un finale necessario per il ricambio dell'umanità». Sosteneva di aver curato 30.000, forse 50.000 pazienti. Veronesi diceva che la morte è un fatto naturale, è parte del disegno biologico della natura che prevede il nascere, il riprodursi e il morire; così è per ogni organismo vivente. Se si ha consapevolezza di questo principio, la morte si affronta con più serenità. Egli sosteneva anche che la scienza non si occupa dell'immortalità, ma di durate della vita in buona salute. Sosteneva: «Una vita intensa dilata il tempo che, per sua natura, scorre incurante e inesorabilmente. Siamo noi che dobbiamo adattarci e trovare, nella durata della nostra vita, la miglior capacità di esprimerci. Il cervello è il direttore d'orchestra: non svilupparlo, allenarlo, espanderlo, renderlo sempre più vivace, significa sprecare la componente più straordinaria del nostro corpo». Alla domanda su cosa avrebbe voluto fosse scritto sulla sua lapide, egli rispose: «Qui giace un uomo che ha contribuito al controllo del male del secolo».

Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, ho il privilegio di ricordare Umberto Veronesi in quest'Aula, la stessa dove nella scorsa legislatura lo abbiamo visto al lavoro. Mi piace ricordarlo dicendo che se ne è andato un grande scienziato, un grande medico; se ne è andato un uomo dal tratto affabile, disponibile, rassicurante; ma se ne è andato anche un italiano rispettato nel mondo, un precursore dei tempi, un uomo dalla forte passione civile e politica, un pioniere della moderna oncologia. Mi permetto di dire, comunque la si pensi, che se ne è andato un vero liberale, nel senso più profondo del termine. Ciò che Umberto Veronesi ha fatto, soprattutto nel campo della senologia oncologica, possiamo dire che ha cambiato la storia della medicina e ha restituito la speranza e il sorriso a tante donne. Battendosi in favore dell'umanizzazione delle cure, ha messo per sempre al centro il paziente e così ha rivoluzionato anche la chirurgia del tumore al seno, proponendo per primo interventi non invasivi grazie a lui che più di vent'anni fa la mastectomia totale ha lasciato il posto

che ha segnato l'inizio di una vera e propria era della nostra medicina. Le donne, anche quelle che non hanno avuto un'esperienza diretta della malattia, sanno a cosa mi riferisco. Umberto Veronesi ci ha insegnato a non avere più paura della malattia e ad avere fiducia nella scienza. non si morirà più di tumore, si morirà con il tumore. E tutti noi sappiamo quanto questa fiducia, ancora oggi troppo spesso messa a dura prova da nuovi forti e pericolosi rigurgiti oscurantisti, costituisca una fiammella fondamentale da mantenere sempre accesa, purché sempre saldata saldata e ancorata tenacemente ai valori della ricerca e della scienza. L'attenzione al paziente, l'umanizzazione delle terapie, la fiducia nel metodo scientifico e la capacità di guardare sempre al futuro con fiducia e razionalità sono valori che Veronesi ha trasmesso alla comunità scientifica italiana e internazionale e che oggi sono un patrimonio consolidato del nostro sistema sanitario e dell'intero mondo della ricerca. Grazie anche al suo generoso impegno e alle sue straordinarie intuizioni scientifiche, l'impegno oggi profuso per il cancro ci consente di non considerare questa malattia come incurabile: sempre più italiani sanno che i tumori possono oggi essere sconfitti con terapie efficaci e con la diagnosi precoce, ma che possono anche essere prevenuti deriva il suo impegno in molteplici campagne di sensibilizzazione per far comprendere agli italiani l'importanza degli stili di vita corretti e della sana e corretta alimentazione. Credo che umanizzazione e innovazione al tempo stesso possano definirsi la cifra distintiva dell'impegno dello scienziato, dell'uomo, del ricercatore Umberto Veronesi,

da poco Ministro della salute nel Governo Amato e io ero consigliere della Regione Puglia. Mi esponeva con passione e con grande semplicità il progetto di cui era promotore con Renzo Piano per ridisegnare e migliorare la qualità degli ospedali italiani, tutti costruiti in una logica e con una prospettiva nuova e diversa, secondo i principi della edilizia dipartimentalizzata. Dal connubio con Renzo Piano e altri architetti nacque un decalogo sul quale si sono basati molti dei progetti dei nuovi ospedali italiani costruiti da allora fino a oggi, e che dovrebbe costituire ancora oggi una pietra miliare per la costruzione dei prossimi: umanizzazione, urbanità, interattività, socialità, organizzazione, appropriatezza, affidabilità, innovazione, ricerca, formazione. Ho voluto ricordarli perché credo che, specialmente oggi, in presenza delle difficoltà in cui si dibatte il Servizio sanitario nazionale, tra sostenibilità, universalità ed equità, si avverte l'esigenza di garantire di più e meglio il diritto alla salute, anche attingendo al cospicuo lascito di proposte, di idee, e metodi di lavoro che Umberto Veronesi ci lascia. Credo proprio che, nel nostro non semplice compito di legislatori, la lezione e l'eredità di Umberto Veronesi, in quella stessa logica che lei, Presidente, poc'anzi ha ricordato facendo riferimento alla figura di questo illustre collega e scienziato, riferita alla scienza e alla ragione, miscelate in un equilibrio straordinario, rappresentino un'importante eredità sotto il profilo del percorso percorso e della prospettiva per costruire un orizzonte che ci dia maggiori certezze e minori preoccupazioni. Il modo migliore per onorare la sua memoria è quello di onorare questi impegni.

quelli che trattano di grandi cose testimoniano, che gloria dona al prode uomo una seconda vita, ciò è a dire, che dopo la sua morte, la nominanza che rimane di sue buone opere mostra ch'egli sia ancora in vita». io credo che Umberto Veronesi resterà per sempre in vita anche se noi sapremo, con tenacia, con impegno e con onestà intellettuale, restituire non solo dignità alla politica ma anche dare un senso pragmatico e operativo al nostro impegno quotidiano di legislatori. È questo l'auspicio che mi fa concludere questo pensiero, con il quale rivolgo una testimonianza sentita di cordoglio e vicinanza, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti, alla famiglia, alla comunità scientifica e a tutta questa Assemblea che ha avuto l'onore di annoverarlo tra i suoi più

Signor Presidente, a nome del Governo mi associo alle tante parole che sono state dette dai colleghi in quest'Assemblea in onore di Umberto Veronesi.

a testimonianza di quanto questo Paese sia grato a suo padre per ciò che ha dato a tutti noi. Umberto Veronesi era un intellettuale sociale, un socialista liberale, uno scienziato che si è battuto sempre - spesso controcorrente - per le persone, per i diritti di scelta delle persone, in particolare e anche nei momenti più complicati della vita. La dignità delle persone era il faro che illuminava, insieme alla libertà delle stesse. Ha abbattuto muri sociali e muri civili e, soprattutto, il grande muro del pregiudizio. Un grande medico, che si è impegnato oltre se stesso per il diritto alla vita e per la qualità della vita delle donne. Esprimeva un concetto dell'etica non come dogma, ma come ricerca perpetua. A sproposito spesso si parla del bene comune. Lui era un operaio del bene comune. Lo ricorderemo per lo spirito libero e impegnato, la cui laicità lo portava ad essere lieve avanguardia civile. In politica ha trasmesso quei valori, ha aiutato ad innovare regole e ad ampliare concetti e la politica lo onorerà se saprà evitare di volgere lo sguardo all'indietro, alimentando invece il futuro di diritti che strappano il paravento del rifiuto dell'altro diverso da noi, il paravento della paura, il paravento dell'indifferenza. uno dei non molti che quando interveniva in televisione richiamava attenzione, per cui si poteva di dire di lui e a lui: «Non ti ho visto ma ti ho ascoltato». Con questo ricordo e con un animo intenso vorrei dire al figlio Alberto che le condoglianze del Governo e del Paese sono un atto molto sentito e molto dovuto.

È un passaggio fondamentale, per ricostruire quel patto di fiducia tra pazienti e operatori sanitari, ma anche tra operatori sanitari e organizzazione. È una pagina nuova e importante che sostituisce la brutta storia degli ultimi anni, caratterizzati dalla medicina difensiva, causata da un innumerevole aumento di ricorsi che hanno creato una situazione di difficoltà nel rapporto medico-paziente rapporto medico-paziente e una discussione e decisioni non sempre all'altezza della sfida sulla questione dell'appropriatezza della cura. Sappiamo che il rapporto medico-paziente è, per molti aspetti, l'elemento fondamentale della buona cura; cura; se il rapporto è di sfiducia è lì che vengono deluse le aspettative. Ma è, invece, proprio qui, nel rapporto medico-paziente, che si può e si deve fare moltissimo per risolvere questo problema e questa legge lo fa. D'altra parte, ristabilire la fiducia del paziente nel medico, ma anche del medico nel paziente è un aspetto troppo sottovalutato; è invece un elemento cruciale per la genesi della paura alla base della medicina difensiva. ricostruire la fiducia tra medico e paziente, serve la disponibilità di entrambi, medici e pazienti, e questa legge pone le basi. Ma serve anche che le amministrazioni della sanità, le Regioni, le ASL, ma anche lo stesso Governo tengano presente che il tempo dedicato al paziente è elemento inscindibile per l'appropriatezza della cura e non tempo perso. Naturalmente questo ha a che fare con l'organizzazione sanitaria. Dicevo che la medicina difensiva è divenuta negli ultimi anni una delle problematiche di crescente impatto sulle politiche sanitarie, essendo essa strettamente collegata al tema della sicurezza della cura, nonché degli eventi avversi e delle eventuali responsabilità professionali.

sia dall'aumento delle aspettative, dalla pressione dei *mass media*, da mutamenti intervenuti nell'ambito del rapporto medico-paziente. Ma un altro elemento importante è stato, nel corso del tempo, l'evoluzione giuridica del concetto e della funzione della responsabilità sanitaria rispetto a comportamenti ed eventi avversi riferibili a possibili errori. Ma anche su questo aspetto, sulla necessità di fare chiarezza e di definire

Guardate, questo provvedimento - va detto in modo molto forte - volta pagina: innova e risponde pienamente alle aspettative dei professionisti sanitari e dei cittadini. Lo stesso titolo tiene insieme, in un *unicum* inscindibile, la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli operatori sanitari. Abbiamo fatto una scelta importante in Senato: abbiamo modificato il titolo e abbiamo appunto tenuto insieme in modo inscindibile sicurezza e responsabilità, perché, se l'avessimo indirizzato, com'era nel titolo precedente, alla sola responsabilità professionale, sarebbe potuto apparire, nell'inconscio e nel messaggio esterno, anche come un atto di medicina difensiva. Mentre, insieme alla sicurezza delle cure, il primo obiettivo

D'altra parte, il tema della sicurezza delle cure è oggi una delle sfide più importanti per il futuro della sanità del mondo occidentale, anche di quella italiana. Ciò è in relazione sia alla limitatezza delle risorse che all'invecchiamento della popolazione, ma anche ad una medicina sempre più complessa per numero di patologie e di strumenti clinico-diagnostici disponibili. Quindi è davvero necessario puntare sul controllo e sul contenimento del rischio, se vogliamo ridurre il contenzioso giudiziario e i costi dei risarcimenti.

parli in modo chiaro della sicurezza delle cure. Sto pensando appunto all'articolo 1, dove viene specificato che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività. davvero importante, che al comma 2 dell'articolo 1 si evidenzia ancora di più, perché appunto si afferma che la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, e l'utilizzo appropriato

dell'articolo 1, che alle attività di prevenzione del rischio concorre tutto il personale, compresi i liberi professionisti che ivi operano in regime di convenzione, questo aspetto non riguarda solo il pubblico, ma tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Un altro aspetto importante è all'articolo 2, che assegna al difensore civico regionale le funzioni di garante per la salute. Altrettanto importante è l'istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi e sugli eventi avversi, nonché sul contenzioso, e trasmette tutto questo semestralmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale (anche questo è un passaggio importante), all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche nella sanità. Tale osservatorio ha un compito importante, quello di individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione dei rischi sanitari, nonché il monitoraggio delle buone pratiche. Anche qui voglio sottolineare l'importanza dell'obiettivo dei sistemi di segnalazione, che naturalmente, oltre a consentire una misurazione del fenomeno, costituiscono un elemento importante, cioè un volano di cambiamento organizzativo e culturale, favorendo tra l'altro un approccio all'errore non finalizzato o almeno non solo finalizzato

non può essere del tutto eliminato, è altresì vero che l'organizzazione deve tendere a creare le condizioni affinché l'errore sia per quanto possibile evitabile e nel contempo creare un ambiente in cui i professionisti possano esprimere al meglio professionalità e competenze. Dobbiamo essere consapevoli che l'organizzazione rappresenta un fondamentale strumento di promozione della salute. Occorre lavorare quindi affinché si accantonino i modelli di intervento individuali e informali, a vantaggio di modalità formali e condivise. Guardate che tale approccio organizzativo, che sta dentro la legge, perché ne è una conseguenza, ne è una conseguenza, consente di fare una cosa importante: incrementare l'affidabilità del sistema e ricollocare in una giusta dimensione le aspettative del paziente, nonché le scelte dei professionisti, conferendo tra l'altro una nuova valenza, più partecipata e trasparente, alla relazione medico-paziente. medico-paziente. Davvero i percorsi organizzativo-assistenziali consentono di superare quell'etica della autoreferenzialità che ancora oggi caratterizza alcuni ambiti professionali.

assegnate all'Osservatorio previsto all'articolo 3 vi è quella della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario. Questo è un punto importante. Tra l'altro, sulla formazione era già intervenuta la legge di stabilità dell'anno scorso, con il famoso comma 539

Noi sappiamo che, ai fini della appropriatezza nonché della sicurezza e qualità delle cure, la formazione gioca un ruolo strategicamente rilevante e che è da realizzarsi sia nella fase accademica che, in modo continuativo, per l'intera attività professionale. La formazione deve consentire a tutti i professionisti di affrontare il cambiamento in sanità, che non è mai fine a se stesso, non solo per i cambiamenti tecnologici ma perché cambiano le malattie e cambiano le richieste dei cittadini. Occorre rafforzare gli aspetti del lavoro in *team*, ma anche dell'autoriflessione e della valutazione dell'attività e degli strumenti per migliorarla. La formazione, oltre che puntare a un cambiamento culturale e valoriale, deve garantire ai professionisti l'acquisizione della flessibilità necessaria per gestire l'innovazione e i cambiamenti dentro contesti di cura sempre più complessi, che chiamano in campo una capacità relazionale e un'interdisciplinarietà. Ultimo aspetto che vado a sottolineare è l'importante

Avendone parlato con tanti, la convinzione è che con questa legge il sistema sanitario, i professionisti e i cittadini potranno ritrovare la centralità: della propria professionalità, da un lato, e del diritto ad avere cure appropriate, dall'altro. E ciò non potrà che avere due effetti: il risparmio delle risorse e il miglioramento della cura.

e ringrazio vivamente i colleghi e gli Uffici per il lavoro svolto. Spero, comunque, che vengano accolti anche ulteriori emendamenti migliorativi. Il Paese ha bisogno di un aggiornato quadro normativo di riferimento in una materia che, per le dimensioni del contenzioso che la caratterizza, ha assunto grande rilevanza: per le relative problematiche di medicina difensiva si calcolano circa dieci miliardi l'anno, circa il 20 per cento della spesa sanitaria, e vi è inoltre un grande problema per l'allungamento delle liste di attesa. Come si evince dai dati emersi dal lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta della XVI legislatura sugli errori in campo sanitario, il 99,1 per cento della cause si conclude con l'assoluzione. Ma questo significa che, quasi sempre, il medico subisce un danno alla propria carriera e alla propria immagine professionale. Credo che questo testo consegua un giusto equilibrio tra medico e paziente. Un medico che non sia timoroso di agire, un paziente che non sia debole nei confronti del medico. Il diritto di curare liberamente e il diritto di essere curati al meglio. È pertanto destituita da ogni fondamento l'idea che alcuni si sono fatti che il testo in esame sia sbilanciato in favore dei professionisti; bensì va a costruire un nuovo rapporto medico-paziente che mi auguro serva a riaffermare un reciproco rapporto di fiducia e di vera alleanza terapeutica, necessario per entrambi. È un rapporto che si sta affievolendo anche grazie ai *media,* che approfittano dei rari casi di malasanità in Italia, non dovuti al nostro sistema sanitario - un'eccellenza nel mondo - ma a singoli casi, per svilire un'intera categoria di sanitari, che, soprattutto oggi, in carenza di fondi, operano spesso in situazioni drammatiche. È però, a mio avviso, necessario garantire con chiarezza un sistema adeguato del rischio clinico rispetto alle responsabilità dei singoli attori. Penso si debba ulteriormente migliorare e chiarire il tema delle linee guida, che non devono essere retroattive e devono essere molto chiare, anche se da medico posso dire che le linee guida a volte non sono seguite pedissequamente, ma servono soprattutto per quelle persone che hanno meno esperienza. Vi faccio un esempio brevissimo: in neonatologia le linee guida dicono che un grave prematuro, intorno ai 700 grammi di peso e con determinati parametri vitali, deve essere lasciato a sé e vedere se sia in grado di sopravvivere. Al di sopra degli 800 grammi sono invece le cure della terapia intensiva. Ora, come può un medico di esperienza, di fronte a un prematuro di 700 o di 680 grammi, con parametri che dimostrano la sua vitalità e la sua vivacità, abbandonarlo e magari accanirsi terapeuticamente - cosa che non succede - su un prematuro di 850 grammi che dimostra chiaramente che potrà essere solo un vegetale?

Ritengo che la previsione di un'azione diretta del presunto danneggiato nei confronti dell'operatore non risolverà completamente il problema della medicina difensiva e necessiterà di polizze onerose soprattutto per ortopedici, ginecologi e neurologi. Spero anche in un ripensamento in merito alla differenziazione tra la lettura extracontrattuale della responsabilità dei professionisti e quella contrattuale delle strutture, nonché, in merito alla disciplina dell'azione di rivalsa, meritano un'ulteriore riflessione le conseguenze degli accordi extragiudiziali conclusi dalle aziende con i pazienti

dei costi delle assicurazioni, soprattutto per i giovani medici. Spero comunque che con l'approvazione di questa legge si possa finalmente allineare l'Italia agli ordinamenti europei più avanzati in tema di responsabilità dei professionisti sanitari. *(Applausi

e un ringraziamento importante anche al Governo, nella persona del sottosegretario De Filippo, ma anche al ministro della giustizia Orlando, alle Commissioni e al lavoro importante, non solo di grande collaborazione, ma di approfondimento, che è stato svolto al Senato con le Commissioni che di questa norma

il confronto nel Paese. Non si contano neanche le iniziative promosse dai parlamentari, che si sono svolte in in tantissime città del Paese e che hanno visto coinvolti, in una discussione puntuale e precisa, i soggetti interessati al provvedimento

un percorso importante, che non solo ci ha aiutato a capire e a comprendere, in una materia così complessa e difficile, quali dovessero essere le giuste scelte, che dessero davvero il segno di una riforma complessiva, quale quella che oggi discutiamo in questa Aula e di cui il Paese aveva bisogno.

la legge che ha come primo obiettivo quello di ricostruire il tessuto sfilacciato della fiducia e

Ci tenevo a sottolineare l'aspetto importante della filosofia che ha accompagnato il provvedimento.

un importante risparmio economico per il Servizio sanitario nazionale. Non sto qui ad articolare le ragioni per le quali penso questo perché sono state abbondantemente illustrate in questi due giorni.

sono tante anche in questo campo. Con un Servizio sanitario nazionale modello in Europa per diritti e garanzie, questo era l'aspetto che ci poneva all'ultimo posto per

le professioni sanitarie, che è anche sotto il profilo psicologico, un elemento fondamentale della riuscita degli interventi di cura,

soprattutto per superare gli aspetti che hanno riguardato il percorso giuridico. Sappiamo quanto importante sia stato il confronto

una uniformità di pensiero sulla necessità di approvare questa normativa. Io penso che la discussione sugli emendamenti, che avverrà a partire da

importante una relazione di fiducia e di rispetto reciproco tra il sistema nazionale della sanità e i cittadini italiani.

presenziato al dibattito. Vorrei ringraziarli perché nei loro interventi hanno ulteriormente chiarito il senso e la portata di questo provvedimento, condividendo quello che nella mia relazione introduttiva al dibattito avevo segnalato. credo che la mia replica si possa tranquillamente limitare ad alcuni aspetti che nel corso del dibattito hanno registrato qualche preoccupazione, se non qualche differenziazione.

noi sappiamo da tempo (ed è consolidato nella letteratura e nell'orientamento tecnico-scientifico e professionale), che le linee guida sono delle raccomandazioni, degli orientamenti, degli strumenti di aiuto alle decisioni, proprio perché anche lo sviluppo della medicina da questo punto di vista ci fa comprendere quanto sia complicato, su situazioni

Questo è già noto. Diventava un passaggio un po' più delicato una volta trasferito nella norma penale o nella norma civile, che noi sappiamo essere inquadrabile sotto forma di norme cautelari.

modo e come venissero definite perché possano assurgere alle caratteristiche di norme cautelari. Questa è stata una preoccupazione, ma è anche vero, devo dire,

non deve necessariamente attenersi alle linee guida quando queste non siano coerenti e adeguate al caso concreto, intendendo per caso concreto non un anonimo, un astratto paziente di un *trial* ma quel paziente, con la sua storia clinica, con la sua complessità clinica, umana, relazionale e quant'altro oppure alle condizioni oggettive in cui si opera: la disponibilità di diagnostica, di strumenti, di organizzazione e così via. Quindi direi che la magistratura ha perfettamente inquadrato, da questo punto di vista, l'ambito delle linee guida. Non a caso nel testo, rispetto al decreto Balduzzi,

di costruire un sistema di produzione di linee guida che avesse una sua solidità. Intendiamoci, parliamo di solidità dei soggetti che propongono le linee guida e dei soggetti che tali linee guida devono assumere, trasferendole nelle pratiche professionali, nelle attività quotidiane e nelle logiche di efficacia e costo-efficacia che sono strumenti di *governance* del sistema di tutela della salute. Naturalmente, preoccuparsi anche della qualificazione metodologica con cui vengono costruite le linee guida. Non stiamo parlando di cose astratte

di coinvolgimento di soggetti, di gruppi scientifici e di comunità scientifiche, come avviene in altri Paesi ma lo scopo è dare un sistema certo, affidabile e trasparente cui riferire le scelte, cui riferire i comportamenti, cui riferire le condotte professionali e io aggiungerei anche le condotte organizzative e gestionali delle organizzazioni. La seconda questione è un po' più delicata e riguarda la responsabilità civile delle strutture e dei professionisti.

contenute in una relazione dei lavori della Commissione nazionale istituita dal ministro della salute Lorenzin sul tema della medicina difensiva e della responsabilità professionale.

della struttura sanitaria. Uno degli elementi del dibattito è stato proprio la distinzione fra la responsabilità contrattuale della struttura e e la responsabilità extracontrattuale degli esercenti le professioni sanitarie che operano dentro le strutture. Voglio solo ricordare il testo stabilisce che i professionisti che assumono direttamente un'obbligazione contrattuale con il paziente mantengono la responsabilità per l'obbligazione, cioè una responsabilità contrattuale. Naturalmente, Naturalmente, la Commissione era composta da giudici presieduti dal presidente del consiglio nazionale forense, esperti di medicina legale, clinici e funzionari del Ministero. Nella «È appena il caso di aggiungere che il modello italiano, nella configurazione che è andata via via assumendo, differiva dalla gran parte dei modelli degli altri ordinamenti dei Paesi membri dell'Unione europea, in cui,

Quei modelli distinguono inoltre in modo netto le posizioni della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione medica, perché perché tengono conto del fatto che la struttura sanitaria offre un servizio articolato, comprensivo di ospitalità, servizi, della fornitura di farmaci e di strumenti medici, di terapie principali e collaterali, ed è, pubblica o privata che sia, convenzionata o meno, un'impresa, come intesa nel linguaggio del diritto comunitario, mentre l'esercente la professione sanitaria svolge un'attività intellettuale. Ai fini della reazione dell'ordinamento, in caso di danni al paziente, si giustifica, dunque, un diverso trattamento dell'una e dell'altro». Io aggiungerei, oltre alle cose della struttura, che

è un inciso che è risultato molto confuso nell'orientamento. Ad ogni modo «volendo anche definire univocamente e conclusivamente le problematiche inerenti la natura e l'ambito della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria ritiene che il testo dell'articolo 3 possa essere migliorato, statuendo che l'esercente, dipendente o convenzionato, risponde in sede civile esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2043 del codice civile,

da questa esigenza, da questa scelta di separare i due profili di responsabilità. testo abbiamo più volte specificato che laddove l'esercente, anche se lavora in una struttura, operi in ragione di un contratto assunto con il paziente, la sua responsabilità resta contrattuale. Abbiamo fatto lunghe audizioni in Commissione su questa materia; sono venuti i giudici del tribunale di Milano e quelli di Cassazione, chi pro e chi contro, e chi contro, ma questo è l'ambito in cui si muove la logica della riforma sul piano della responsabilità civile.

preliminare, sollevata dal senatore D'Ambrosio Lettieri, credo sia un problema vero. Il problema è che bisogna cambiare il codice di procedura penale (mi sembra l'articolo 550 del codice di procedura penale), comprendendo anche l'imputazione per lesioni tra le cause che possono avviare la procedura. Non siamo ancora arrivati a quel grado di elaborazione, di confronto anche molto positivo con tutte le componenti (magistrati, Ministero della giustizia) per questo; ritengo pertanto che il richiamo possa trovare una sua memoria nel testo anche con delle soluzioni possibili, magari in un successivo provvedimento che guardi alla riforma del codice di procedura penale.

La novità sta nel fatto che diventa una procedura obbligatoria nei casi di responsabilità. Non credo si pongano problemi

quando parliamo di costi e di velocità ci riferiamo a diritti dei cittadini, perché l'accesso ad un risarcimento rapido ed equo è innanzitutto un interesse del cittadino. Il problema si pone perché la nostra legislazione

L'osservazione che viene fatta è che come la legge sopprime il ricorso a questi altri strumenti potrebbe essere ingiustificato o ingeneroso, e credo che una qualche ragione in questo ragionamento ci sia, ricordando soprattutto che l'istituto della conciliazione di fatto ha cominciato a funzionare tre anni fa,

che considera gli obblighi per le imprese private, quali sono le assicurazioni, delle violazioni della libera circolazione dei servizi e della concorrenza.

Ringrazio ancora l'Assemblea e spero che la mia replica, se non altro, possa avere dato soddisfazione alle ragioni degli altri, che legittimamente possono mantenere.

voglio innanzi tutto - devo dire con grande franchezza - non formalmente ringraziare il senatore Bianco per il lavoro che, anche nella replica, ha dimostrato essere certosino, competente.

che, ancora una volta, insieme dimostrano, per la mia esperienza, quanto può essere serio e fruttuoso il nostro lavoro quando è totalmente ripiegato sul merito dei problemi. Grazie veramente per la emblematicità di questa circostanza e di questa esperienza su questo provvedimento che, insieme a voi, ho potuto vivere nei lunghi mesi di discussione. sarà molto lunga; mi sentirei di fare soltanto alcune riflessioni a commento di un dibattito molto importante. Negli ultimi anni si è registrato un considerevole incremento del contenzioso in ambito sanitario. Ciò ha comportato innanzi tutto un ricorso crescente alla cosiddetta medicina difensiva che, attraverso le molteplici prestazioni diagnostiche e terapeutiche, anche non necessarie o, al contrario, in molte circostanze con la rinuncia a interventi necessari, ma che potevano apparire ad alto rischio, ha determinato una pluralità di conseguenze negative per la salute stessa dei cittadini, e sicuramente un aumento stimato - ma non puntualmente calcolato - della spesa sanitaria.

Sia Agenas che alcune organizzazioni mediche, per fare solo brevissimi riferimenti, hanno svolto indagini sulla materia e in alcuni casi hanno evidenziato che si raggiunge anche il 10 di prestazioni sanitarie che potrebbero essere considerate come medicina difensiva: dai farmaci alle visite, dagli esami di laboratorio agli esami strumentali, fino a ricoveri non necessari. Ovviamente, al di là dei dati che sono comunque da giudicare con rigore e con attenzione - e uno degli elementi che il disegno di legge prova ad affrontare è esattamente la ricostruzione

che occorre affrontare in maniera sistematica, come prevede molto puntualmente il provvedimento all'esame di quest'Assemblea. Un altro aspetto particolarmente preoccupante è quello dell'esodo dalle specializzazioni maggiormente esposte maggiormente esposte a rischi. Presumibilmente nei prossimi anni potrebbe verificarsi la necessità di ricorrere a medici provenienti da altri Paesi su branche specialistiche che sono rifiutate da studiosi e medici italiani per il rischio che contengono nelle loro prospettive professionali. Occorre, infine, ricordare che molti professionisti sanitari nell'attuale sistema non riescono ad ottenere un'adeguata copertura assicurativa sul mercato per i costi eccessivamente alti delle polizze e per un mercato assicurativo del nostro Paese che

addirittura extraeuropei, con tutte le implicazioni di competenza e di difficoltà che in queste alleanze assicurative si possono strutturare rispetto al sistema sanitario italiano. L'orizzonte che il legislatore aveva davanti era, quindi, particolarmente scoraggiante e ha richiesto un lavoro veramente complicato. Nella consapevolezza di queste problematiche, negli ultimi tre anni, in particolare, il Ministero è stato fortemente impegnato sul tema della responsabilità professionale sanitaria,

alle criticità derivanti dalla rigida applicazione dei principi generali sanciti dal codice civile e dal codice penale in materia di responsabilità professionale nell'esercizio di un'attività ad alto rischio come per sua natura è quella medica. convertito in legge, aveva altresì previsto che, con decreto del Presidente della Repubblica, fossero disciplinate le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, nonché la costituzione di un apposito fondo per garantire un'idonea copertura assicurativa a chi non fosse riuscito a trovarla sul mercato. L'*iter* complicato di quel provvedimento ne segnala proprio la difficoltà applicativa: si è rivelato sicuramente un *iter* molto lungo per la complessità di questa materia,

Tuttavia, nonostante lo scenario abbastanza difficile, dopo aver effettuato numerosissimi approfondimenti, con*dossier* e documenti (vi è una bibliografia e una documentazione

che i tempi fossero maturi per un intervento organico in materia. Lo scorso anno presso il Ministero è stata pertanto costituita, con un decreto dello stesso Ministro, un'apposita commissione - i cui lavori sono stati citati da ultimo dal senatore Bianco secondo me di alto livello, presieduta da un esperto come il professor Guido Alpa e composta da tutte le professionalità che hanno in qualche modo funzioni, esperienze o implicazioni sulla materia (giuristi, magistrati, avvocati, medici, esperti di *risk management*), per elaborare una proposta finalizzata a sciogliere i tanti nodi del problema. La commissione ha lavorato a ritmi sorprendentemente serrati e già prima dell'estate del 2015 ha consegnato al Ministro una relazione, che è stata successivamente inviata

del quale occorre da un lato assicurare ai professionisti la giusta serenità nell'esercizio della propria attività e dall'altro garantire ai cittadini incorsi in casi di *malpractice* il giusto risarcimento per i danni subiti, è apparso indispensabile procedere esattamente a questo lavoro, anche di tipo culturale. Infatti la relazione del professor Alpa, citata dal senatore Bianco, inquadra la questione in un contesto scientifico, giuridico e bibliografico di rango europeo, dove il tema della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale, con fondamenti giuridici o addirittura filosofici riferiti in quella relazione, ci dà il senso di una traiettoria sulla quale abbiamo voluto fortemente interagire con il Parlamento. Vorrei sintetizzare in altri tre o quattro punti questioni che sono nella sistematicità di questo provvedimento. Il disegno di legge all'esame del Parlamento affronta a tutto tondo il problema delle responsabilità dei professionisti sanitari e in generale i temi connessi a questa questione. *In primis* segnalo che, con l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, collegato ai centri per la gestione del rischio clinico di livello regionale,

Insomma, si prefigura con l'elaborazione di questi dati, cosa non trascurabile nel provvedimento in esame, un vero e proprio sistema nazionale sia sul *risk management*, ma anche sulla prevenzione, che sostanzialmente potrà potrà produrre nel tempo, secondo noi, un grandissimo cambiamento di sistema. Anche la tempistica, i luoghi, le procedure e le metodiche che sono più sottoposte a rischio clinico di eventi avversi potranno essere di per sé un grandissimo patrimonio per attivare meccanismi e metodiche di prevenzione molto più efficaci. Io non trascuro questa parte della norma, che implementa esattamente questo sistema di dati in maniera molto più puntuale, nella trasparenza e nell'efficacia che il provvedimento prevede. Sulla sicurezza delle cure occorre evidenziare che alcune disposizioni in materia di governo del rischio clinico, originariamente contenute nel disegno di legge, sono già state inserite nella legge di stabilità al comma 538. In particolare, secondo quanto previsto da queste ultime disposizioni, le Regioni dovranno disporre che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, quindi su scala aziendale, su scala ospedaliera, su scala regionale e su scala nazionale. In questa piramide sostanziale sta - secondo me - una delle architetture molto efficaci che il sistema sanitario potrà realizzare nei prossimi anni. Come si vede, l'ampiezza del provvedimento ha obiettivi di riorganizzazione complessiva.

sulla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, si dettano, in quelle parti del provvedimento, disposizioni in materia di responsabilità civile e penale dei professionisti sanitari. In considerazione proprio del diverso rapporto giuridico che si instaura tra il paziente e il medico, a seconda che quest'ultimo agisca quale libero professionista o quale dipendente di una struttura, si prevede la responsabilità a doppio binario. Segnalo che si avrà una riduzione

Vengono poi previsti ulteriori limiti alla responsabilità per colpa grave, ove il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, sulla quale questione ha redatto una scheda molto puntuale, da ultimo, il senatore Bianco. Le linee guida sono un *discrimen* fondamentale della responsabilità. Il sistema che si intende implementare con questa legge sulla parte relativa alle linee guida è secondo noi molto efficace. Prevede, innanzitutto, una istruttoria e un filtro importante su chi le scrive, su quali sono i soggetti autorizzati e su come vengono implementati i sistemi che, all'interno del Servizio nazionale, in in una azione tecnico-scientifica, che non può che essere un *work in progress* - come sono notoriamente le linee guida - dovranno essere in condizione di aggiornare efficacemente e con grande trasparenza. l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie. Si introduce tale obbligo per tutte le strutture, sia pubbliche che private. È introdotta l'azione di rivalsa da parte delle aziende nei confronti dei propri dipendenti. Anche in questo caso, vi sono norme molto chiare. Ancora, vi è il fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Si demanda a un regolamento l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per i casi di *malpractice*, volto a risarcire le vittime nel caso in cui non si possa provvedere con le assicurazioni. al tentativo obbligatorio di conciliazione, si introduce l'obbligo di esperire preliminarmente ai giudizi civili un tentativo obbligatorio di conciliazione, con le osservazioni sulla mediazione, che il Governo condivide, segnalate nel dibattito non solo dal senatore Bianco ma anche dal senatore D'Ambrosio Lettieri. una più trasparente compilazione degli elenchi dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti. Si prevede che le consulenze tecniche nei giudizi civili e penali siano affidate non solo al medico legale, ma anche a uno specialista nella disciplina oggetto di contenzioso. Insomma,

e prioritariamente a consolidare i nuovi diritti per i pazienti/utenti, che avranno più sedi e migliori procedure per difendersi (dal difensore civico, ai procedimenti stragiudiziali, ai tribunali) con azioni dirette, facilitate dalla nuova normativa - non trascuro questa parte decisiva del provvedimento - e altresì un quadro più sicuro per i professionisti della sanità, che potranno svolgere il loro lavoro con più tranquillità e, quindi, con più efficacia e sostenibilità nel sistema sanitario italiano.

Il sistema sanitario italiano ha bisogno veramente di questo provvedimento e il clima che si respira in quest'Aula è davvero incoraggiante e di grande livello.

Lo faccio perché, dopo le parole del relatore e soprattutto dopo quelle del Governo, non voglio rompere l'incantesimo, nel senso che mi sembra giusto,

consapevole, autonomo, libero informato e responsabile. Temo che, attesa l'assenza dei colleghi per ovvi motivi, stiamo proseguendo

con riferimento alla pacificazione del rapporto tra operatore sanitario e utente e tra medico e paziente, la stella polare di questo provvedimento, sulla quale abbiamo costruito un ragionamento e abbiamo tentato anche di alimentare in modo corretto e proficuo il nostro dibattito, si concentra proprio attorno ai percorsi di sicurezza delle cure. Credo che si consegua in modo efficace il principio di sicurezza delle cure anche attraverso

dell'informazione e della trasmissione dei dati sui rischi e sugli eventi avversi alla Regione di appartenenza. Per la verità, gli aspetti inerenti l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso alle prestazioni sanitarie, e quindi, di conseguenza,

puntuale, preciso e che non lasci spazio a equivoci, perché non venga tradita la volontà del legislatore, quando a valle questo provvedimento dovrà essere

ci sia coerenza tra le previsioni dell'articolo 1 e quello dell'articolo 2 in relazione alla circolarità delle informazioni. Colleghi, all'articolo 2 è espressamente previsto che in ogni Regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario Il compito di questo Centro è di raccogliere i dati regionali sui rischi e trasmetterli all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che è richiamato all'articolo 3. Poi, successivamente, all'articolo 3 si dettaglia più precisamente quale sia il compito dell'Osservatorio nazionale e quali sono le finalità

del rischio, adottando idonee misure, finalizzate al buon governo della sanità, attraverso la patrimonializzazione di queste informazioni.

anche attraverso una buona lettura, prima, e un buono utilizzo, dopo, dei dati che si riferiscono allo *status* in cui versa la sanità, in cui si vengono a erogare le prestazioni sanitarie, con l'individuazione dei punti di criticità: si tratta del principio della prevenzione non soltanto della malattia, ma anche delle inappropriatezze e delle *malpractice*, che generalmente sono motivo di distorsione di un sistema che, con con grande fatica, ma anche con grande impegno, stiamo tentando di spingere in una zona di maggiore chiarezza.

si orienta anche l'emendamento 2.203 che, per così dire, è legato all'articolo 1

ha avuto la possibilità di esplicarsi nella libertà e nella possibilità di approfondire le buone pratiche

risponde lo Stato e, solo in via di rivalsa, il magistrato. Grosso modo in alcune parti avete tentato di ricostruire questo schema.

che in quella occasione le buone pratiche hanno portato a un risultato positivo anche al di là delle linee guida o non previsto dalle linee guida, in quel caso la punibilità è esclusa. Allora, non c'è bisogno di parlare di imperizia o di raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate alla specificità del caso concreto. Bisogna dire che la punibilità è esclusa nel momento in cui sono rispettate le linea guide oppure se, con accertamento tecnico, il giudice verifica che le buone pratiche hanno portato a un risultato positivo per l'ammalato.

Oggi i componenti della commissione d'inchiesta della Regione Toscana ci hanno chiesto espressamente di prenderci carico

dopo aver svolto per due consigliature due commissioni di indagine e dopo aver ascoltato le diverse vittime della cooperativa, a chiederci di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare e di spingere il Governo a un commissariamento della cooperativa

Ci sono vittime che ancora oggi hanno difficoltà a dormire; ci sono vittime che non hanno sopportato quello che hanno subito e si sono tolte la vita. Noi, in qualità di parlamentari italiani, abbiamo il dovere di di mettere la parola «fine» come parte politica a questa vicenda. La magistratura ha fatto il suo, ma noi dobbiamo prenderci le responsabilità di quel "sistema Forteto" che non ha funzionato. E, quindi, chiedo a tutti voi di sottoscrivere

un caffè! Oggi io e il collega Stefano Lucidi ne abbiamo ampiamente parlato e ragionato proprio davanti a un caffè. Per un caffè noi stiamo vendendo la democrazia o, comunque, una buona parte di democrazia che i nostri Padri costituenti ci hanno dato. Questo è il costo che si andrebbe presuntivamente a risparmiare sulle indennità che non verrebbero più erogate ai senatori. Ma è un caffè. Per un caffè noi vendiamo parti di sovranità popolare. Il sistema partitico negli anni ha capito che, lasciando al cittadino la possibilità di votare, stava perdendo consensi. Quindi ha cominciato innanzitutto a creare le liste bloccate; poi, nel momento in cui, nell'ultima legislatura, ha capito addirittura che le liste bloccate non gli bastavano più, ha deciso di farsi una Camera tutta sua, tutta sua, il Senato; tutta sua, la Camera alta; tutta sua, perché i cittadini non voteranno mai più il Senato della Repubblica. Questa è una riduzione delle prerogative popolari

che vogliono proporci ha dei limiti, e il limite è quello di non votare mai più il Senato. Io credo, signora Presidente, che per un caffè non è possibile vendersi la democrazia che i nostri Padri costituenti ci hanno dato, e ce l'hanno data anche con il sangue.